del 19 dicembre 2013 e in una seduta del febbraio 2014 si parlò di una vicenda che riguardava la mia persona e alcuni colleghi, contestando alcuni fatti, chiesero anche - ma questo può accadere - le mie dimissioni. Io svolsi un intervento in cui spiegai dettagliatamente le circostanze di una vicenda giudiziaria che mi riguardava e l'Assemblea ebbe la compiacenza di ascoltare con grande rispetto e attenzione

all'Assemblea del Senato, perché nella sede giudiziaria ieri è stata riconosciuta con una sentenza di assoluzione l'insussistenza del fatto. Vorrei che questo rimanesse agli atti.

dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali», collegato alla manovra di finanza pubblica. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi

comma 2-*bis* del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, osserva che il termine del 31 gennaio indicato dall'articolo 7, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 196 del 2009, per la presentazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, non è stato rispettato, in quanto il disegno di legge in titolo risulta presentato alla Presidenza del Senato il 16 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, può considerarsi dì carattere ordinatorio. Rileva, altresì, che le disposizioni del disegno di legge risultano, nel loro complesso, funzionali al miglioramento dell'efficienza del settore del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo, nonché al riordino della normativa in materia di attività culturali, conformemente alla Nota di aggiornamento e al Documento di economia e finanza 2015, e che esse appaiono, inoltre, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come sancito dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità». Tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge collegato n. 2287, ai sensi dell' articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del provvedimento in questione non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.

quella dei minori sottratti a livello internazionale è una situazione non ancora esplosa all'attenzione né dell'opinione pubblica né dei *media*, ma neanche della politica e delle istituzioni.

Quel che è certo è che il fenomeno è in crescita, anche a causa dell'aumento di relazioni tra persone di nazionalità diverse; unioni spesso caratterizzate da un'elevata conflittualità dovuta anche alle differenze socio-culturali e religiose che inducono, nei casi più estremi, alla sottrazione del figlio da parte di uno dei due genitori. Ho partecipato nelle settimane e nei mesi scorsi a incontri e convegni in cui erano presenti molti genitori, i cui figli sono stati sottratti. Ho ascoltato le loro parole di dolore - un dolore che definirei agghiacciante - con cui hanno raccontato l'odissea vissuta nel tentativo di avere notizie del figlio, e anche solo di poterci parlare. persone che spesso si scontrano con lungaggini burocratiche, con un diritto che quasi sempre si ferma ai confini del proprio Stato; persone che hanno avuto anche una sentenza esecutiva, che non si riesce però a fare attuare. sono persone sfinite anche economicamente, perché nella ricerca del figlio investono tutto: tempo, risorse e spesso lasciano il proprio lavoro. A tal proposito sottolineo, rispetto anche a quanto chiesto nella mozione,

al gratuito patrocinio per tutte le domande presentate ai sensi del capo III della Convezione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori. E questo è davvero un risultato importante e auspichiamo che rapidamente l'Atto venga approvato. La sottrazione internazionale di minori è un tema molto delicato da affrontare sotto molti punti di vista: sotto i profili giuridico, sociale e culturale. È un tema che chiama tutti noi a delle responsabilità, Parlamento e Governo. E non dimentichiamo che è un tema che coinvolge, ma anche sconvolge, la vita degli adulti, ma soprattutto quella dei minori: bambini e bambine improvvisamente sradicati dalla propria vita quotidiana, dai propri affetti familiari e amicali. È un tema che necessita di tener conto dei principi ampiamente tutelati dalle convenzioni internazionali, a partire da quella dell'Aja. Mi riferisco al diritto di avere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambi i genitori anche dopo la separazione e il divorzio, così come al diritto di preservare la propria identità, compresa la nazionalità, il nome e le proprie relazioni familiari, nonché il diritto di essere tutelato contro illegittimi trasferimenti all'estero. Ad oggi l'unico strumento utilizzato è la Convenzione dell'Aja, ratificata da 93 Paesi. È l'unico strumento giuridico internazionale cogente cui è possibile ricorrere per i casi di sottrazione internazionale, ma anche per la regolamentazione del diritto di visita con Paesi non appartenenti all'Unione europea. Va detto, però, che le procedure previste da tale Convenzione non trovano identica e uniforme applicazione in tutti gli Stati, poiché l'attuazione dipende dalle singole normative di recepimento. Infatti, tale strumento convenzionale è di per sé debole per tre specifici punti: per i tempi insostenibili dell'*iter* giudiziario (mediamente tre gradi di giudizio); di giudizio); per le frequenti interpretazioni strumentali dell'articolo 13 della Convenzione da parte degli organi di giustizia del Paese verso cui il minore è sottratto. Infatti, l'articolo 13 prevede le eccezioni al rientro del minore sottratto, come - ad esempio -

di molti Paesi di religione islamica e di diversi dell'estremo Oriente. Ad oggi sono troppi i casi di contrasto giurisprudenziale tra Paesi che alimentano le dispute tra genitori e producono ulteriori danni allo sviluppo di quel minore già messo alla prova dalla sottrazione e, quindi, dalla rottura dei propri legami. Infatti, anche quando ci sono sentenze dei tribunali, esistono serie difficoltà a farle eseguire e ciò da parte sia dei tribunali italiani che di quelli dei Paesi in cui i minori sono trattenuti. la Convenzione dell'Aja stabilisca la competenza del giudice del Paese in cui il minore risiede, rimangono davvero troppe le difficoltà ad eseguire le sentenze approvate. Conseguentemente a tali difficoltà, nostro esame si propongono alcune decisioni su cui si sollecita l'azione del Governo: in merito alla prima, stante la difficoltà di applicazione e la grande difficoltà di fare eseguire le sentenze, si propongono trattati bilaterali promossi dal Ministero degli affari esteri, sia con gli Stati aderenti alla Convenzione ma anche con gli altri, perché riteniamo che la snellezza degli accordi tra due soli Paesi determini un criterio di reciprocità a tutto vantaggio di una rapida soluzione dei singoli casi, nell'interesse superiore del bambino. Si propone poi di agire in ambito europeo e internazionale affinché siano previste sanzioni verso i Paesi inadempienti agli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa e siano anche studiate e messe in atto misure diplomatiche e politiche adeguate al fine di indurre tali Stati a un atteggiamento più collaborativo. Questa scelta, però, ha bisogno che l'Europa parli con una sola voce, per cui si sollecita il Governo italiano a porre in ambito europeo la questione dell'avvio di un'azione politica per giungere a un unico diritto di famiglia a livello europeo. Altra questione cruciale su cui chiediamo l'impegno del Governo è la necessità di sveltire e semplificare le procedure amministrative e giudiziarie, anche attraverso un maggiore raccordo istituzionale, poiché la molteplicità delle competenze istituzionali allunga i tempi e il tempo fa la differenza quando un bambino scompare, quando lo si rintraccia e quando si può rientrare a relazionarsi con lui. Noi oggi abbiamo tre Ministeri competenti in materia: gli esteri, la giustizia e gli interni. Sappiamo che il Ministero di giustizia, che interviene tramite l'Autorità centrale centrale istituita presso il dipartimento di giustizia minorile, si attiva per i casi riguardanti Paesi nei quali è in vigore la Convenzione dell'Aja, mentre il Ministero degli affari esteri ha competenza per i casi che non hanno avuto esecuzione tramite la Convenzione dell'Aja e per i casi che coinvolgono Stati non aderenti alla Convenzione di Bruxelles. Altresì il Ministero degli affari esteri, nei casi di sottrazione, può fornire, attraverso i propri consolati, assistenza al genitore e al bambino italiani e, ove opportuno, sostenere le procedure avviate dai legali. Infatti, il console generale ha funzione di giudice tutelare per i minori italiani residenti nel territorio di sua competenza. Uno degli impegni richiesti con questa mozione è diramare a tutte le ambasciate italiane nel mondo un protocollo d'intesa sulle iniziative da intraprendere in caso di sottrazione, come ad esempio l'accompagnamento del genitore che tenti di esercitare il suo diritto di visita perché, ad oggi, vi è un atteggiamento un atteggiamento completamente diverso da ambasciata ad ambasciata. L'ultimo Ministero competente è quello degli interni, che deve vigilare le frontiere e gli aeroporti al fine di evitare la sottrazione. Anche questa attività è resa più complicata, insieme alle altre, per il fatto che in Italia il nostro ordinamento non prevede uno specifico reato di sottrazione di minore. Mentre in gran parte dei Paesi occidentali tale fattispecie esiste e viene considerata reato di grave allarme sociale, in Italia è normata è normata dall'articolo 574-*bis* del codice penale, e cioè all'interno della sezione codicistica inerente ai delitti contro la famiglia e non invece, come dovrebbe, come reato contro la persona e la libertà personale. Infatti, il bene giuridico protetto non è la libertà del minore, ma la sola potestà dell'altro genitore, di quattro anni come massimo edittale della pena determina l'inapplicabilità dei principali e più efficaci mezzi di protezione e di ricerca delle persone. Parlo delle intercettazioni telefoniche e ambientali, ma anche delle misure cautelari e custodiali. Sono quindi tre i Ministeri coinvolti ed è evidente che tale molteplicità di competenze allunga l'*iter*. Per questo il cuore della proposta è istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato interministeriale diretto da commissari straordinari.

Successivamente a separazioni, divorzi e quant'altro, nascono le dispute e i minori si trovano in una contesa che non appartiene loro, in quanto gli stessi dovrebbero avere

nel senso che nel matrimonio misto è molto difficile far convivere culture davvero distanti, a patto che non vi sia un accordo ferreo tra i due genitori. Far vivere i propri figli in questo Paese significa adottare tutte le regole e le garanzie che il sistema occidentale offre. Se a un certo punto qualcuno dei due coniugi decide in modo diverso, nascono le problematiche che noi tentiamo oggi di far arrivare come monito al Governo, perché normative, convenzioni internazionali e azioni di su quanto la mozione della Lega Nord chiede al Governo.

un nuovo articolo del codice penale che disciplini una nuova fattispecie: sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori. E, proprio per dare massima efficacia, bisogna che questo introducendo articolo nel codice sia anche procedibile d'ufficio. Qualora nei confronti del minore sottratto vi siano non soltanto intenzioni

e che in questo caso non si possano nemmeno applicare le attenuanti previste dagli articoli 62 e 62-*bis* del codice penale. Sottoponiamo inoltre al Governo la necessità di costituire un *pool* di magistrati esperti,

o addirittura di bambini che dall'estero vengono portati illecitamente qui in Italia e sottratti alle loro famiglie di origine.

per i genitori inizia il grande calvario. Come spiegava molto bene prima la collega Mattesini, improvvisamente questi bambini, sottratti - lo ripeto - illecitamente, non hanno più punti di riferimento e diventano invisibili anche anche per le amministrazioni statali. Perché dicevo prima che il fenomeno è conosciuto e ha radici antiche?

la Convenzione europea di Strasburgo, la Convenzione dell'ONU di New York del 1989, oltre naturalmente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950. Eppure, ancora a oggi il fenomeno non è assolutamente circoscritto. In Italia cosa accade? Vi sono diverse competenze:

del Ministero degli affari esteri abbiniamo anche la responsabilità delle ambasciate, ossia quegli addentellati nel mondo che rappresentano il nostro Stato e che spesso e volentieri si trovano a dover fare da cuscinetto tra gli interessi del minore e del familiare a cui è stato illecitamente sottratto e lo Stato nel quale l'ambasciata

aprire una parentesi su un'esperienza che ho vissuto in prima persona. Quando in questo Parlamento abbiamo affrontato il problema delle persone scomparse - anche in tal caso le competenze erano di diversi Ministeri la cosa più naturale che ci è venuta da chiedere e da mettere in campo è che uno si prendesse la responsabilità di fare da coordinatore. Se un genitore che richiede di essere ascoltato deve peregrinare tra il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero di giustizia e scrivere *e-mail* all'ambasciata di appartenenza,

un Ministro, un Sottosegretario, un funzionario sia il punto di collegamento tra i tre Ministeri e le ambasciate di riferimento sia soprattutto l'interfaccia responsabile e accogliente per quei genitori disperati. Chiediamo anche che in Italia l'inasprimento dell'articolo 574-*bis* sia veramente effettivo e che questo sia un reato: è un reato

tutelati e di autotutelarsi. Quindi i più grandi, i più responsabili e il nostro Governo devono saperli tutelare. Chiediamo di aiutare quei familiari con un fondo *ad hoc*

Chiediamo che i rapporti bilaterali che L'Aja richiedeva e che ha messo in atto siano ancora più stringenti

tutte le ambasciate, relativamente all'accoglimento delle istanze di questi genitori, ma anche risposte concrete di cuscinetto, come dicevo prima. intensifichiamo i controlli alle nostre frontiere. Quando un genitore esce dal perimetro italiano con un figlio, cerchiamo di capire esattamente se è totalmente lecito o se si sta nascondendo un illecito.

vorrei porre in evidenza anzitutto come il fenomeno delle sottrazioni internazionali di minori sia in continuo aumento e, con il passare del tempo, stia diventando sempre più grave e preoccupante. È stato più volte posto all'attenzione, ma ancora non riesce a trovare una soluzione adeguata e soddisfacente. Tale fenomeno è dovuto a diversi fattori come, appunto, il numero sempre maggiore di convivenze e matrimoni tra persone di diversa nazionalità, che sono il risultato anche dell'incremento dei flussi migratori degli ultimi decenni. Alla base si riscontrano molto spesso contrasti dovuti ai diversi costumi e usanze, diversità religiose, che portano a soluzioni estreme da parte di uno dei due genitori con la sottrazione del figlio per trasferirlo con sé nel proprio Paese di origine. È bene chiarire come per sottrazione internazionale di minori si intende il caso in cui un minore che possiede la residenza abituale in un determinato Stato è stato condotto in un altro Stato, senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale e, quindi, anche il diritto di determinare il luogo di residenza abituale del minore. Viene equiparato, inoltre, alla sottrazione anche il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, senza il consenso del genitore o di un altro soggetto titolare dell'affidamento. Stiamo parlando di un vero e proprio sequestro di persona, a cui si aggiunge il fatto che il soggetto vittima di questo atto è un minore, con tutte le implicazioni che ad esso derivano dalla sua situazione di ridotta difesa data appunto la minore età. Gli effetti sono devastanti non solo per la serenità del minore sottratto, ma anche in quanto procurano enormi preoccupazioni e sofferenze al genitore che si vede sottratto il proprio figlio. Ciò che deve essere tutelato è proprio il diritto per i figli ad avere rapporti stabili e duraturi con entrambi i genitori - nel caso di separazioni o divorzi - per far sì che possano crescere che possano crescere serenamente e con l'affetto del padre e della madre ai quali è riconosciuto il diritto di genitorialità. In materia di sottrazioni internazionali esistono diversi strumenti giuridici per la tutela del minore a livello internazionale, anche se questi non sono ancora in vigore in tutti gli Stati. La Convenzione dell'Aja del 1980, ratificata dall'ordinamento italiano con la legge n. 64 del 1994, a cui aderiscono finora 93 Paesi, ha come obiettivo il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale. Attualmente la Convenzione rappresenta l'unico strumento giuridico internazionale a cui è possibile ricorrere per salvaguardare l'interesse del minore. Tuttavia, è da notare che non vi è uniformità di applicazione delle procedure previste dalla Convenzione in tutti gli Stati, la cui attuazione dipende invece dalle singole normative interne. La Convenzione è valida solo per i Paesi contraenti (europei ed extraeuropei). Per quanto riguarda l'attuazione operativa della Convenzione, essa è demandata alle cosiddette autorità centrali di ciascuno Stato contraente, incaricate di perseguire le previsioni della Convenzione e di collaborare tra loro al fine di garantire la sua attuazione. In Italia, il ruolo di autorità centrale è affidato al Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile, al cui interno è stato costituito l'ufficio II - autorità centrali convenzionali. Si tratta appunto della localizzazione del minore illegalmente trasferito o trattenuto, al fine di assicurare che avvenga la consegna volontaria o agevolare una composizione amichevole; lo scambio di informazioni relative alla situazione sociale del minore; l'avvio delle procedure giudiziarie o amministrative, volte al rientro del minore o, nel caso, a consentire il diritto di visita; organizzare la predisposizione, a livello amministrativo, delle misure necessarie per garantire il rientro del minore in condizioni di sicurezza. Sempre a livello internazionale possiamo citare ulteriori strumenti giuridici a tutela del minore sottratto. Vi è per l'appunto il regolamento n. 2201 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003, chiamato anche regolamento Bruxelles II-*bis*, avente l'obiettivo di istituire uno spazio comune europeo in materia di diritto di famiglia. Il suddetto regolamento si integra con la Convenzione dell'Aja in materia di sottrazione di minori e prevede la competenza del giudice del Paese dove il minore risiedeva prime della sottrazione e l'esecutività delle decisioni emesse dal giudice competente provviste del certificato *standard*, cioè del titolo Inoltre, regola la materia la Convenzione ONU di New York del 1989 sui diritti dell'infanzia, ratificata con la legge n. 176 del 1991. Si segnalano l'articolo 3, che evidenzia il principio del superiore interesse del bambino; l'articolo 8, volto alla preservazione dell'identità del minore, compresi la sua nazionalità, nome e le sue relazioni familiari; articoli 9 e 10, riferiti ai rapporti personali e diretti con entrambi i genitori; infine, l'articolo 11 per la tutela del minore contro trasferimenti illegittimi all'estero. Tale Convenzione, insieme ai suoi protocolli opzionali, rappresenta lo strumento più completo per la tutela dei diritti dell'infanzia. Ulteriori strumenti giuridici sono la Convenzione europea di Lussemburgo del 1980 e quella di Strasburgo del 1996, nonché la Convenzione europea per la del 1950, che è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea e il cui articolo 8, in tema di diritto al rispetto della vita privata e familiare, è stato più volte utilizzato nelle controversie per minori contesi. A fronte di un quadro normativo internazionale così ampio, ad oggi il fenomeno delle sottrazioni internazionali dei minori non ha ancora trovato una decisiva soluzione. In Italia possiamo notare una scarsa tutela offerta dall'articolo 574-*bis* del codice penale, dovuta alla collocazione della medesima norma tra i delitti contro la famiglia e non contro la persona o la libertà individuale. Allo stesso modo è previsto un massima di pena, pari a quattro anni di

lo strumento si è dimostrato non sufficiente nel risolvere in maniera favorevole i numerosi casi di sottrazione di minori che ormai si trascinano da anni. anni. Il Gruppo Forza Italia esprime la necessità che venga istituita un'unità di crisi presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o un organismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per esaminare e valutare le denunce di minori sottratti illecitamente o trattenuti all'estero e di predisporre, in accordo con il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno, le azioni necessarie per favorire il rientro in Italia del minore sottratto. Rileviamo come sia necessario un nuovo strumento operativo che sia in grado di con maggiore incisività con i Governi di Stati esteri per risolvere in maniera definitiva le problematiche relative alle sottrazioni di minori.

Presidente, colleghi, è una consuetudine parlamentare alquanto discutibile considerare strumenti di indirizzo politico talmente rilevanti come le mozioni alla stregua di atti marginali. Le mozioni vengono inserite e tolte in un calendario dei lavori indirizzato verso ciò che il Governo e la maggioranza ritengono essere la priorità del Paese, senza considerare quali siano realmente, come in questa occasione. La mozione che oggi mi appresto a illustrare, che verrà discussa congiuntamente con le mozioni presentate dagli altri Gruppi parlamentari, infatti i minori, nonché il loro diritto ad essere protetti e non essere privati di uno o di entrambi i genitori viventi e non pericolosi per la loro incolumità psichica o fisica. Dopo averlo più volte visto inserito in calendario e poi tolto, oggi finalmente affrontiamo il tema della sottrazione internazionale dei minori. un fenomeno in continua crescita, perché sono in aumento i matrimoni e le unioni tra persone di diversi Paesi e culture. Tuttavia, non esistono relazioni semestrali sul numero delle persone scomparse che permettano di fotografare la situazione nel suo complesso e con la precisione che meriterebbe. Pochi giorni fa stata pubblicata la relazione semestrale, dopo un'assenza di anni. Considerando i dati pubblicati nell'agosto dello scorso anno, sarebbero 610 i minori dei quali si sono perse le tracce, mentre risultavano essere 341 nell'anno precedente i casi di minori sottratti da parte di un genitore o altro congiunto. I diversi soggetti istituzionali competenti nel nostro Paese in materia sembrano condizionati negativamente, nell'efficacia e rapidità della loro azione preventiva, da un approccio riduttivo e meramente casistico del problema. Tale orientamento dovrebbe invece lasciar posto posto ad un metodo del tutto differente, riconoscendo che al caso di un bambino sottratto - fosse anche uno

i reati di sottrazione internazionale dei minori. Vi sono competenze riconosciute in capo al Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, alla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, alle ambasciate italiane nel mondo e, per ultimi ma non per importanza, alla Commissione per le adozioni internazionali e al Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Oltre alla frammentarietà e diversificazione delle competenze tra i vari organismi testé richiamati, il vero anello debole, in materia di sottrazione di minori, è rappresentato nel nostro Paese dalla legislazione. L'attuale articolo 574-*bis* del codice penale offre, infatti, una tutela inefficace in questi casi perché inserisce il reato di sottrazione di minore tra le fattispecie dei delitti contro la famiglia e non contro la persona o la libertà individuale, come di fatto è, perché un minore non sceglie volontariamente di interrompere i rapporti con un genitore e l'ambiente parentale formato da nonni, zii e cugini, cui è legato affettivamente. Nell'ottica punitiva di tale abuso, l'individuazione in quattro anni della pena massima comminata a chiunque sottragga il minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale risulta essere insufficiente e poco poco scoraggiante per chi ha intenzione di mettere in atto simili azioni deprecabili e, soprattutto, impedisce l'utilizzo di alcuni efficaci mezzi di prova come le intercettazioni ambientali e telefoniche, che sono utilissime in questi casi. Tale quadro è ulteriormente inficiato dalla poca efficacia degli accordi internazionali tuttora in vigore in materia. Penso, in primo luogo, alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia ratificata nel nostro ordinamento con la legge n. 176 del 1991, nella quale sono sanciti principi fondamentali per la tutela del diritto del minore a preservare l'identità, la nazionalità e le relazioni familiari, nonché di intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori e a essere tutelato contro gli illegittimi trasferimenti all'estero.

il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale. Tuttavia, la medesima Convenzione non risulta essere applicata adeguatamente. Fatte queste dovute premesse e venendo all'analisi nel merito del testo, con questa mozione a mia prima firma si vuole impegnare il Governo ad assicurare un maggiore coordinamento organizzativo dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia di sottrazione internazionale dei minori sia nell'ottica della prevenzione che in quella del maggiore supporto investigativo, finanziario e psicologico alle persone coinvolte; a sostenere, per quanto di competenza, opportune iniziative di carattere normativo, volte a inasprire il quadro sanzionatorio in materia di sottrazione internazionale dei minori, nonché a rafforzare la fattispecie di reato anche attraverso l'inserimento della stessa nell'ambito dei delitti contro la persona e la liberta personale; a promuovere, mediante il Ministero degli affari esteri, la stipula di accordi bilaterali con gli Stati firmatari e non firmatari della Convenzione dell'Aja, introdotta nel nostro ordinamento come avevo detto precedentemente, in modo da favorire, nell'esclusivo interesse del minore, la rapida soluzione

per la definizione di sanzioni concrete a carico di quei Paesi che non adempiono agli obblighi derivanti dalle Convenzioni, cagionando un danno fisico e psicologico soprattutto in capo ai minori, ad elaborare e indirizzare alle rappresentanze diplomatiche italiane nel mondo atti dettagliati di indirizzo politico, nei quali sia fissato un termine perentorio di due settimane, entro il quale ambasciate o consolati devono far pervenire una risposta ai tribunali italiani che hanno disposto il rientro del minore nel Paese d'origine.

dove, grazie allo spirito collaborativo instauratosi tra il procuratore capo Cappelleri e la polizia giudiziaria, è stato risolto più dell'80 per cento dei casi,

alcun altro tipo di interesse che sia del tutto estraneo alla impellente, trasparente e doverosa esigenza di dare risposte concrete ai genitori vittime di sottrazioni internazionali di minori.

e questo *trend* è in netta crescita. Ogni anno più di 310.000 nuove coppie di nazionalità diversa si sposano e altri 140.000 matrimoni si concludono con separazioni o divorzi. Quando si parla di sottrazione internazionale di minori si fa infatti riferimento alla fattispecie nella quale, in seguito alla rottura di un rapporto genitoriale misto, uno dei due genitori decida di fare ritorno al Paese di origine, portando con sé la prole. Questo è un evento traumatico per chi lo subisce, una violenza intrafamiliare che turba ogni possibile equilibrio e genera danni importanti nel processo di crescita e di formazione della personalità del bambino o dell'adolescente. La disciplina della sottrazione internazionale di minori prende spunto dalla Convenzione dell'Aja del 1980, ratificata da 93 Paesi, e poi dal regolamento di Bruxelles II-*bis*.

ad oggi senza una sua base giuridica. In pochi sono a conoscenza della genesi di questo ruolo, che nasce addirittura nel 1987, su iniziativa

Nel tempo l'ufficio del mediatore ha operato *de facto* come una finestra aperta al pubblico dei genitori separati, senza però mai dotarsi di una base giuridica, né di una solida struttura amministrativa. Il che ne ha impoverito notevolmente le competenze nonostante l'enorme potenziale sia sul profilo del contributo legislativo, che sull'assistenza ai minori. Questo servizio, nonostante le enormi potenzialità, è assolutamente inadeguato così come strutturato, soprattutto perché convertitosi, nei costumi del Parlamento, in un accessorio del Vice Presidente di turno, senza alcuna continuità e struttura amministrativa e dunque senza alcuna garanzia per i cittadini, nonostante la sensibilità dei casi trattati. L'altro punto è quello della necessità di un migliore coordinamento tra le due figure cardine di tutta la materia: le autorità centrali da una parte e lo stesso ufficio del mediatore del In effetti questo ufficio fornisce ai genitori un'assistenza tesa alla ricerca di una via alternativa all'azione giudiziaria, che è potenzialmente lesiva per gli interessi del minore. Questo lo dovrebbe fare (anzi, lo farebbe) attraverso una conciliazione o una risoluzione alternativa per risolvere questa controversia. Inoltre, potrebbe svolgere un importante ruolo diplomatico nel coordinamento di queste procedure, che tutti avete detto che sono complesse, tra l'autorità e gli Stati membri che ne sono coinvolti. È l'autorità centrale a raccogliere le denunce dei vari soggetti colpiti ed è proprio da questa che l'ufficio del mediatore europeo ottiene molte delle informazioni utili per svolgere il proprio compito. Questo stesso ufficio ha difficoltà di comunicazione con i genitori, oltre a ingenti ritardi nelle indagini procedurali. Pertanto auspico soprattutto una maggiore attenzione da parte degli operatori proprio sulle tempistiche, dato che gli interessi in gioco sono altissimi ed è molto difficile che questi siano risarcibili in forma pecuniaria come un qualsiasi danno di tipo civile. civile. Il nostro compito è quindi quello di puntare sulla prevenzione. Dobbiamo imporre alla Commissione di elaborare un *vademecum* valido per tutti gli Stati membri e tradotto in tutte le lingue dell'Unione europea, dove si parli di affido condiviso, di sottrazione internazionale di minori, ma dove si parli anche di diritti e doveri dei genitori e soprattutto dei diritti dei figli. Certo, questa informazione non risolverà tutti i casi ma sarà utile per accendere qualche lampadina, far sorgere qualche dubbio e quindi, magari, qualche problema si potrà anche evitare. Come al solito, è meglio prevenire che combattere. Altro problema è la scarsa informazione tra i professionisti, in particolare tra quelli più giovani. Il cliente va guidato nelle scelte da chi esercita la professione, con criteri ovviamente giuridici, e non etici, visto che spesso quel cliente che abbiamo seduto davanti non ha chiaro l'interesse del minore. La funzione preventiva dell'avvocato serve a guarire quella che io chiamo una disfunzione cerebrale, ovvero quell'atteggiamento che spesso porta il genitore a volere a tutti i costi allontanare la prole dall'ex *partner*

è molto più comune l'ostinazione attraverso forme legali, verso l'altro coniuge. C'è come una rivalsa; una ferita e un'offesa che io devo guarire punendo l'altro coniuge. È importante anche un elenco di comportamenti che l'avvocato può consigliare al proprio cliente al fine di prevenire eventuali e spiacevoli fattispecie di sottrazione internazionale del minore. luogo, si può chiedere al giudice del tribunale che ordini alla questura una revoca dell'autorizzazione all'espatrio. Si può segnalare alla rappresentanza consolare di un altro Stato il proprio dissenso rispetto alla concessione del visto. Si può pretendere, nel caso di un minore che deve recarsi all'estero per vacanza, la sottoscrizione di un impegno al rientro (ad esempio in Italia) davanti all'autorità consolare del Paese in questione. Si può chiedere di vietare l'espatrio senza il consenso di entrambi i genitori. Si può chiedere di far riconoscere allo Stato di appartenenza dell'altro genitore il provvedimento che vieta l'espatrio o contenere tempi di permanenza per problemi specifici. Ricordiamoci tutti, alla fine, che i minori sono passati negli ultimi anni dall'essere, anziché un mero oggetto di sottrazione, oggetto di protezione, fino a divenire veri e propri titolari di diritti; ecco allora la necessità di ascolto durante i procedimenti, tesi al conseguimento del cosiddetto *best interest* del minore. Su queste controversie giudiziarie non ci si contende una casa, un anello, un conto corrente, ma ci si contende un ragazzo, a volte un bambino. Quindi, si discute come se fossero oggetti di scambio, ma sono costretti, loro malgrado, a vivere in una duplice sofferenza: da una parte, la perdita dell'altro genitore e la necessità di vivere in una situazione di semiclandestinità; dall'altra, un conflitto permanente tra il desiderio di ricomporre questo nucleo familiare - o quantomeno di riunirsi al genitore lontano - e la necessità di imparare a convivere con il proprio "rapitore", che comunque resta sempre un genitore. Anche quando questi casi vengono risolti al livello giuridico, si incontrano enormi difficoltà a far attuare le sentenze sia nei Paesi italiani sia nei Paesi in cui i minori sono trattenuti. Quindi, l'appello è sulla certezza dell'esecutività delle sentenze e un potenziamento dei poteri dei pubblici ministeri, che ad oggi, ad esempio, non possono richiedere intercettazioni telefoniche o ambientali per questi casi. questi casi. Ci si scontra con ordinamenti giuridici lontani dai nostri, con leggi e procedimenti diversi, e spesso con l'impreparazione dei nostri avvocati nell'affrontare casi che sono regolamentati da un'unica norma, la Convenzione dell'Aja del 1980. Questa è un'ulteriore motivazione per ribadire l'importanza di un'altra figura, quella del mediatore nazionale, affinché sia un punto di riferimento per i cittadini e i genitori che devono affrontare simili difficoltà. Una figura esperta, di ascolto, che possa riportare tali istanze e preoccupazioni ai mediatori internazionali e che rappresenti le famiglie ai tavoli delle trattative dove si possono superare questi contenziosi. Per far ciò è necessaria l'istituzione di uno spazio giuridico europeo armonico e omogeneo. La mancanza di uniformità legislativa, non solo in materia di sottrazione internazionale dei minori, è quindi ritenuta dagli stessi membri del Parlamento europeo una grave mancanza nella vita politica e istituzionale del Continente. Questo oggi è il nostro compito di legislatori: colmare tali carenze nel quadro giuridico. Manca una norma uniforme e completa nelle competenza giurisdizionale atta a coprire tutte le situazioni. In realtà, nella nostra nella nostra mozione chiediamo: di promuovere e potenziare il quadro sanzionatorio mediante l'innalzamento del massimo edittale di pena previsto dall'articolo 574-*bis*.

Salutiamo le studentesse e gli studenti del Liceo «Antonio Rosmini» di Rovereto, in provincia di Trento. Benvenute e benvenuti al Senato.

Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, ne approfitto anch'io per salutare gli allievi del liceo Rosmini di Rovereto, non solo perché provengono dalla mia terra ma anche perché da anni stanno portando avanti un importante progetto di cittadinanza attiva che per fortuna vede coinvolte molte delle nostre scuole. I colleghi che mi hanno preceduto hanno ribadito molti dei dati relativi ai migranti minorenni che risultano scomparsi dopo l'arrivo in Europa, dati che sono allarmanti. Secondo il *report* 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei primi sei mesi del 2015, con gli sbarchi, sono arrivati in Italia 13.320 minori non accompagnati e di questi ben 5.114 risultano irreperibili, scomparsi. Il rischio che questi minorenni finiscano in circuiti illegali, forniscano manovalanza alla criminalità organizzata o siano variamente sfruttati per traffici illeciti non è da sottovalutare. Tale tesi è peraltro avvalorata dalle molteplici associazioni o organizzazioni nazionali ed internazionali che si occupano delle problematiche legate all'infanzia e all'adolescenza. Europol, l'agenzia di sicurezza europea, sostiene che i bambini scomparsi siano stati sequestrati da una struttura criminale per avviarli alla prostituzione o alla schiavitù. Infatti, in Germania e Ungheria, sempre secondo tale agenzia, sono stati arrestati molti criminali legati al traffico di esseri umani, che ora si sarebbe concentrato sulle centinaia di migliaia di disperati giunti in Europa. Secondo l'organizzazione umanitaria Save the children, nel 2015 sono arrivati nel continente 26.000 bambini non accompagnati e, dopo la loro identificazione nel Paese d'arrivo, molti di loro sono scomparsi. «Sono gli Invisibili, non hanno un volto e neppure un nome ma sono giovanissimi, hanno tutti meno di diciotto anni, un'età nella quale i loro coetanei vanno a scuola, fanno i compiti, giocano a pallone con gli amici o nuotano in piscina. Loro, invece, sono vittime di abusi e soprusi». Queste le parole del Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. sulla sorte dei minori che trovano riparo alla stazione Termini di Roma, con molti di loro che, pur di sopravvivere, finiscono per prostituirsi. Per fortuna, lo dobbiamo dire, dei tanti minori giunti nel nostro Paese, non tutti sarebbero finiti nelle mani di criminali, in quanto alcuni sono stati affidati a membri della loro famiglia, ma non si sa dove sono. La sorte dei rifugiati minorenni non accompagnati sta quindi diventando uno degli aspetti problematici della crisi dell'immigrazione e l'Italia sembra essere il Paese che controlla meno i movimenti degli immigrati, anche perché molti dei rifugiati hanno interesse a far perdere le proprie tracce. Il loro obiettivo, infatti, è spostarsi al Nord, in luoghi come la Svezia, che concede asilo ai minori subito dopo averli identificati, o in Gran Bretagna, che ha appena deciso di accogliere più minori dalle zone di guerra.

perché la sparizione di 5.000 minorenni è una questione molto seria e occorre, con la massima urgenza, mettere in campo una politica organica ed adeguatamente finanziata. Nella mia mozione, che è stata sottoscritta anche da molti colleghi che ringrazio, ho chiesto alcuni impegni al Governo alcune urgenti iniziative al fine di rintracciare i bambini, ma soprattutto l'impegno ad avviare un'indagine allo scopo di individuare eventuali organizzazioni criminali che agiscono sul territorio italiano per lo sfruttamento dei migranti minorenni. Anche con le altre mozioni molti impegni sono stati chiesti. Sono convinto che il tema sia veramente veramente molto complesso ma sia anche di grande attualità e drammatico per cui mi auguro che il Governo, al di là dei singoli impegni, prenda a cuore questo problema e trovi il modo per intervenire. In Aula abbiamo parlato spesso del problema dei migranti e anche nel corso dell'ultima relazione del presidente Renzi prima del Consiglio europeo ho avuto modo di ribadire che occorre rivedere l'Accordo di Dublino, occorre snellire e velocizzare le operazioni di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico. Sono problemi sicuramente molto grandi che l'Europa fa molta fatica ad affrontare. Tuttavia io credo credo che soprattutto sull'emergenza relativa ai minori e ai bambini dovremmo mettere in campo un'iniziativa straordinaria e mi auguro che il Governo sappia cogliere questa sollecitazione e trovare assieme a noi il modo per venire incontro a questo dramma nel dramma.

*(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la sottrazione internazionale di minore è un tema particolarmente delicato in quanto si tratta di un terreno ove ove diritto e relazioni umane si intersecano provocando un contemperamento di interessi in gioco estremamente difficile da attuare. La mozione che oggi andiamo a discutere, e che non ho esitato a firmare, espone chiaramente il quadro giuridico e le lacune normative della disciplina, La sottrazione internazionale di minore si verifica quando uno dei genitori decide volontariamente, unilateralmente senza il consenso dell'altro, di sottrarre il figlio con l'intenzione di nasconderlo all'estero e di tenerlo con sé in modo permanente. Un altro caso in cui si verifica la sottrazione del minore è quello in cui al minore stesso venga impedito il rientro nell'abituale stato di residenza dopo un un trasferimento avvenuto per causa legittima, come nel caso di una vacanza, al termine della quale il genitore che ha portato con sé il figlio ne impedisce il rientro nel Paese di residenza abituale. evidente come episodi di tal genere possano arrecare un trauma ai minori che si trovano a dover affrontare il distacco da una delle due figure genitoriali e, nel contempo, il distacco dal contesto di vita nel quale il minore era inserito. La Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176, stabilisce che il minore ha diritto a mantenere una stabile relazione con entrambi i genitori. L'articolo 9 della Convenzione stabilisce, inoltre, il diritto del fanciullo, separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambe le figure le figure genitoriali, a meno che ciò non sia contrario all'interesse del fanciullo stesso. Detto principio è stato ripreso nell'ordinamento italiano, dalla legge n. 54 del 2006, e anche la Corte di cassazione ha specificato che ciò che più rileva è l'interesse del minore a non essere arbitrariamente sottratto al suo ambiente di vita. Il punto focale della questione è rappresentato quindi dall'interesse del minore, che è l'unico a dover emergere ed è l'unico aspetto di cui andrebbe tenuto conto nell'applicazione pratica della normativa. Il diritto del minore alla bigenitorialità, previsto nel nostro ordinamento, che impedisce ad un genitore di privare il figlio dell'altro genitore ed il diritto del minore a non essere sradicato dal centro dei propri affetti ed interessi, ove lo stesso è cresciuto ed ha sempre vissuto, devono essere entrambi tutelati. Lo sradicamento del minore dal proprio ambiente rappresenta infatti un atto di violenza che può causare un gravissimo pregiudizio al benessere psicofisico del minore. Nei casi di sottrazione, come in tutte le decisioni relative ai bambini, deve pertanto essere tutelato in via preminente il superiore interesse del minore a coltivare un rapporto costante e paritetico con entrambi i genitori e a conservare l'ambiente in cui il minore si è integrato e coltiva le relazioni più significative. Quando il minore, abitualmente residente in uno Stato membro, viene illecitamente condotto o trattenuto in altro Stato membro dell'UE da parte dell'altro genitore, si applica la procedura per il ritorno del minore prevista dalle disposizioni della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Come rilevato chiaramente all'interno del testo della mozione, a prima della senatrice Mattesini, sulla quale ci troviamo oggi a discutere, sono tre le principali criticità della normativa attualmente vigente e applicabile: in primo luogo, la lunghezza dell'*iter* giudiziario; in secondo luogo, le frequenti interpretazioni strumentali delle eccezioni al rimpatrio del minore in quanto non è previsto alcun obbligo di dettagliare e dimostrare le presunte «situazioni intollerabili o pericolose» per le quali verrebbe negato il rimpatrio del minore; infine, manca la ratifica di quasi tutti i Paesi di religione islamica e dei Paesi dell'Estremo Oriente, che hanno una cultura, una tradizione, una mentalità e una concezione della posizione della donna e dei minori molto diverse dalle nostre. L'evoluzione in senso multietnico della società civile, i nuovi flussi migratori e la minore solidità delle relazioni familiari rendono sempre più frequente il fenomeno; basti pensare che il totale dei casi nell'anno 2015 ammonta a 211 e di conseguenza è sempre più urgente la necessità di avere una normativa la cui applicazione sia rapida ed efficace e le cui disposizioni siano poste a tutela dell'esclusivo interesse del minore, che è, in tali casi, il soggetto più vulnerabile. Ritengo quindi che debbano essere prese in considerazione e attuate le proposte normative elencate all'interno della mozione, in particolare: la costituzione di un fondo dedicato al gratuito patrocinio per le vittime di

di attribuire maggiori poteri alle ambasciate e, in particolare, maggiore disponibilità per le ambasciate stesse di mezzi e risorse che gli consentano di gestire nel modo più rapido e corretto i rapporti con le autorità estere, fornendo ai genitori che si recano nel Paese ove il minore è stato portato tutta l'assistenza necessaria ad affrontare la situazione. In particolare si dovrebbe creare una sorta di procedura giuridica preferenziale per la gestione di questi casi, ovvero un coordinamento tra strutture, che porti a dei riscontri rapidi; si dovrebbero creare delle figure *ad hoc* come una *task force* legale che possa possa essere dislocata temporaneamente nelle ambasciate per seguire casi particolarmente urgenti o gravi. Nella maggior parte delle sedi diplomatiche non sono infatti presenti figure di esperti legali. I bambini contesi nelle dispute familiari divengono protagonisti di scenari di conflittualità e odio reciproco tra genitori e, nei casi di trasferimento illecito oltre frontiera, vengono improvvisamente privati del rapporto con uno dei due genitori e sradicati dal proprio ambiente sociale, scolastico e geografico. Gli viene negato il diritto alla bigenitorialità e il diritto di mantenere dei rapporti stabili e duraturi con entrambi i genitori. Per evitare ciò è necessario attivarsi e attuare tutte le riforme normative volte a porre l'interesse e il bene del minore al centro delle stesse, al fine di ridurre quanto più possibile traumi e danni irreversibili nella crescita e nello sviluppo del minore.

29.234 persone scomparse: un aumento di 3.170 unità rispetto al 31 dicembre 2014. Secondo l'organizzazione umanitaria Save the children nel 2015 sono arrivati nel Continente 26.000 bambini non accompagnati e dopo la loro identificazione nel Paese d'arrivo molti di loro sono scomparsi. Il quadro allarmante evidenziato da questi dati ci obbliga ad indagare, attraverso un'attenta analisi del fenomeno, quali siano le cause del fallimento dell'attuale impianto normativo posto a tutela dei diritti dell'infanzia. Infatti, se da una parte la normativa internazionale e nazionale pone al centro l'interesse superiore del minore, dall'altra, il costante aumento del fenomeno dimostra che l'attuale assetto giuridico è in definitiva inefficace. Ciò in prima istanza è certamente dovuto dall'assenza di norme internazionali cogenti, che lasciano allo spontaneo recepimento dei singoli Stati l'applicabilità delle norme. Parlo della Convenzione ONU del 1989, che non ha portata immediatamente precettiva e pertanto non può essere fonte di alcun ricorso nel Paese convenuto. Parlo della Convenzione dell'Aja del1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, che è l'unico strumento giuridico internazionale cogente cui è possibile ricorrere per i casi di sottrazione o per la regolamentazione del diritto di visita con

anche questa una convenzione che risulta alquanto debole e che lascia ampio margine di discrezionalità al giudice dello Stato convenuto. È evidente quindi che, per arginare questo fenomeno, è necessario attivarsi per la condivisione delle procedure, arrivando all'istituzione di uno spazio giuridico europeo che sia armonico ed omogeneo e promuovendo la definizione di un unico diritto di famiglia europeo. Allo stesso modo, è importante agire in ambito europeo ed internazionale affinché siano previste sanzioni verso i Paesi inadempienti

quale sia l'autorità giurisdizionale competente ad applicare il proprio diritto sul minore. Vedo che il tempo sta sfumando. Lascerò il testo del mio intervento, affinché sia facendo cenno alla frammentazione di competenze istituzionali, che in Italia sono assegnate, secondo le rispettive competenze, al Ministero della giustizia, alla Direzione generale per gli italiani all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e alle ambasciate italiane nel mondo. Questa frammentazione non produce risultati positivi. È infatti necessario - e quindi appoggio assolutamente quanto è previsto nella mozione a prima firma della Mattesini - assicurare un maggiore coordinamento organizzativo dei diversi soggetti istituzionali competenti e l'elaborazione e la diffusione, a tutte le ambasciate italiane nel mondo, di un protocollo di intesa sulle iniziative da intraprendere in caso di sottrazione di un minore italiano.

alla luce di quello che ho ascoltato, del fatto che il dibattito su questo tema ha incontrato la sensibilità di pressoché tutti i Gruppi presenti in Senato e, soprattutto, per il fatto che i punti sui quali i senatori si sono soffermati sono in gran parte condivisi,

Signora Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi di dire che le mozioni di oggi - finalmente approdate all'esame di quest'Assemblea - rappresentano un segnale di importante presa di coscienza delle istituzioni rispetto ai tragici e complessi fatti denunciati, malgrado i ripetuti e talvolta inevitabili rimandi della calendarizzazione. Il tema trattato resta delicato, doloroso e scomodo per certi versi. Ma oggi, con la mozione a mia prima firma e con le altre depositate in questi mesi, si vuole riservare a questo la giusta rilevanza, non avendo trovato finora l'attenzione giusta nelle agende dell'Esecutivo, sopraffatto per le priorità di ben altra natura. Ma oggi siamo qui perché in territori non tanto lontani dalle nostre case si sta consumando la barbarie per eccellenza, quella che ha come vittime i minori, e dinanzi a questa degenerazione umana uno Stato che si qualifica moderno, democratico e di diritto, non può restare a guardare, limitandosi a manifestazioni per lo più retoriche di condanna. La mozione in esame è figlia dei suoi tempi: sono passati circa tredici mesi dalla sua pubblicazione e dalla presentazione del rapporto del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. del febbraio 2015, lo scenario che avevamo dinanzi era drammatico. Ma la vergognosa situazione che condiziona l'infanzia nei territori di nuova e vecchia crisi, ha subìto un significativo peggioramento, con la terribile impennata dei flussi migratori che si è consumata negli ultimi mesi e l'immagine straziante - ahimè anche strumentalizzata - del piccolo Aylan sulle coste turche ne rappresenta forse l'espressione per eccellenza, in quanto metafora di un fallimento non solo di strategia ma anche di cultura. La cultura del rispetto e del diritto, su cui si è fondata l'Europa moderna, comincia a mostrare le sue falle. Questa mozione vuole affrontare anche questo. Il fatto che questa trattazione avvenga a pochi giorni dalla Pasqua e dalla strage di Lahore in Pakistan assume un valore simbolico ancora più forte. Ricordiamolo insieme: meno di due settimane fa, 72 persone, soprattutto donne e bambini della minoranza cristiana, sono state uccise in un attacco suicida in un parco pubblico. Nell'attentato, rivendicato dai talebani del gruppo Jamatul Ahrar, i *kamikaze* si sarebbero fatti esplodere vicino a delle altalene nel punto centrale del parco. Il simbolo inquietante dell'estremismo religioso accanto ad un gioco innocente in un giorno di festa deve essere l'immagine intorno a cui abbiamo l'obbligo morale di scuotere le coscienze e rimodulare gli strumenti di resistenza ad uno scenario conflittuale oggettivamente mutato. Questi drammi, per certi aspetti ufficializzati all'epoca del citato rapporto ONU, venivano svelati con violenza alla comunità internazionale e il fatto stesso che alla denuncia sia seguito il silenzio conferma il sostanziale fallimento del sistema internazionale. Come qualche altra mozione successiva ha ricordato, vi è stata una risoluzione del Parlamento europeo, che nei fatti resta lettera morta. Il tema dell'infanzia violata viene sempre più spesso schiacciato sotto il peso della presunta maggiore rilevanza di altre questioni nell'area del mediterraneo. Ovviamente questo conferma che dinanzi a tragedie così gravi, figlie di ideologie deviate, l'attenzione della comunità internazionale rischia di essere condizionata dagli equilibri legati alla zona di interesse. Quanto si sta verificando nelle aree di crisi rappresenta una nuova frontiera del terrorismo di matrice islamica, dinanzi al quale sembriamo non avere strumenti di controllo e di lotta adeguati e la cui sistematica persecuzione delle minoranze cristiane rappresenta una delle sfaccettature più atroci. Secondo la World watch list 2016, pubblicata nel gennaio scorso dalla ONG internazionale Porte Aperte, il 2015 è stato l'anno più cruento sul versante della persecuzione dei cristiani. Il numero dei cristiani uccisi nel mondo in ragione della loro appartenenza religiosa è aumentato del 63 per cento. È in atto un vero e proprio olocausto e nessuno sembra volerne parlare. Le principali vittime di questa tragedia sono soprattutto bambini, sistematicamente uccisi, torturati e seviziati dai miliziani dell'ISIS o dai gruppi estremisti attivi nelle varie aree di crisi, in alcuni casi perché i piccoli non vogliono abiurare per convertirsi all'Islam, come testimoniano i tragici fatti di Ninive, in Iraq, del dicembre 2014. L'*escalation* di crudeltà, strategica ed organizzata, degli ultimi mesi è la prova della debolezza di un Occidente narcotizzato. Come non ricordare, in questa sede, le parole di Papa Francesco a proposito della «nostra coscienza insensibile e narcotizzata». Questa radicalizzazione dell'abominio sembra volutamente concentrarsi sui bambini, che sono espressione del futuro e della speranza delle Nazioni e porta con sé un significato che non può essere etichettato come conflitto di civiltà. di qualcosa di più complesso: l'ideologia diventa elemento propulsore di una neoformazione statale che raccoglie nuovi adepti, attingendo a piene mani dal malcontento generale entro cui si collocano le nuove generazioni nei territori di crisi e mostrandosi come unico interlocutore, attivo e deciso, in aree in cui la confusione politica, etnica e di confini rappresenta l'unica certezza. In questo scenario l'esasperazione della violenza, nelle sue forme più atroci e incomprensibili, rappresenta uno strumento esso stesso di comunicazione, attraverso cui mandare all'Occidente un messaggio chiaro di capacità, determinazione e forza. Coinvolgere bambini - siano essi vittime di attentati, schiavi sessuali o *baby* soldati - rappresenta la massima espressione di questo piano strategico, perché toccando i minori si toccano le corde più profonde della coscienza sociale e storica dei Paesi democratici. L'emergenza migranti rappresenta il punto di approdo, tra le altre cose, dell'assenza di una strategia europea. Proprio partendo da questa riflessione, appare chiaro che lo scenario entro cui è stata maturata la mozione in esame è mutato. Come dicevo, lo scenario si è aggravato soprattutto in termini di urgenza nella tutela dell'infanzia violata. Tutto questo impone una revisione dell'approccio e degli strumenti di intervento in generale, ma in particolare della tutela dei minori, soprattutto se si tiene conto che uno dei riflessi più delicati del dramma del terrorismo è rappresentato dall'afflusso in Europa di minori non accompagnati, che è uno degli aspetti più delicati del versante dell'emergenza dei flussi migratori. Secondo i dati Eurostat, nel 2014 i minori non accompagnati sbarcati sulle coste italiane sono stati 7.831 e nei primi due mesi del 2015, dei 7.883 migranti che hanno attraversato il Mediterraneo uno su dieci è minore. Il fenomeno del flusso straordinario di minori non accompagnati sul territorio nazionale non può essere disgiunto dalla trattazione del dramma dell'infanzia nei territori di crisi, trattandosi della sua naturale evoluzione. Dovremmo tener conto di questo anche in un'eventuale mozione unitaria a cui giungere a seguito dell'odierna trattazione. momento, la priorità della comunità internazionale dovrebbe pertanto essere una rinnovata strategia di lotta al terrorismo che parta da strumenti diversi che sappiano adeguarsi all'evoluzione delle strategie di comunicazione ed attuazione del disegno terroristico da parte dei gruppi ferocissimi e che, nel contempo, sia orientata alla stabilizzazione non solo politica, ma anche sociale dei territori sensibili teatro dell'azione sanguinaria di questi gruppi. sede non si discute l'opportunità di intervenire o no militarmente. Voglio che ciò sia ben chiaro, altrimenti l'intera discussione si ridurrebbe alla solita *querelle* tra interventisti e non. Ci attestiamo ben oltre le diatribe geopolitiche e la disgregazione dei confini, dovendoci collocare in una prospettiva di tutela inderogabile dei diritti dei più piccoli e dell'infanzia, che non possono essere immolati sull'altare di alcun altra priorità.

Con la mozione - e con quelle presentate dai colleghi, che sono sostanzialmente affini per elementi evidenziati e per urgenze reclamate - chiediamo una posizione chiara al Governo che si faccia portavoce nelle opportune sedi di passi decisivi e di iniziative valide. In primo luogo, chiediamo di richiamare l'attenzione dei *partner* internazionali, nelle opportune sedi, sulla gravità di quanto verificatosi a danno dei minori nei territori controllati dal califfato islamico dell'ISIS e nelle aree sotto il controllo di Boko Haram in Nigeria, come pure in tutte le zone dove si rilevano derive integraliste di matrice terroristica. Si chiede di elaborare strategie di intervento che vadano a contrastare la degenerazione e la barbarie messa in atto dai gruppi jihadisti a danno, soprattutto, dei minori; a dare impulso, in sede europea ed internazionale, anche attraverso il coinvolgimento attivo di organizzazioni internazionali, ad iniziative volte all'approfondimento di quanto denunciato dall'ONU e alla creazione di canali di aiuto e di supporto all'infanzia nei territori

con il solo scopo di disseminare terrore e piegare un territorio ad un *Diktat*, impone un sollevamento delle coscienze ed un obbligo morale in capo a quei Paesi che ancora hanno l'ambizione di proclamarsi democratici che vada ben oltre i semplici ed infruttuosi proclami di sdegno ma che sappia identificarsi in una strategia valida e condivisa. L'Italia, in ragione delle sue connotazioni geografico-logistiche che la espongono come terra di approdo e di transito dei terroristi - come l'attualità sta evidenziando non può permettersi di indugiare ulteriormente e, di contro, necessita ergersi a portavoce di una iniziativa ferma e risoluta attraverso cui dare forma ed attuazioni a principi inderogabili e inalienabili intorno ai quali abbiamo costruito la nostra democrazia.

noi partiamo da un qualcosa che ci ha letteralmente sconcertato. Mi riferisco al rapporto del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. Il rapporto esamina e definisce la condizione drammatica in cui vivono i bambini e i minori nei territori occupati tanto

il rapporto risale al febbraio del 2015. Sono gli unici dati che abbiamo a disposizione e possiamo pensare che la situazione oggi sia di gran lunga peggiore. Il Comitato descrive il tutto come una tragedia di portata enorme che coinvolge migliaia di minori che si trovano nelle zone di Iraq e Siria e, soprattutto, quei minori che appartengono a gruppi minoritari come cristiani, yazidi e sciiti. Il rapporto denuncia effettivamente molti casi di esecuzione di massa

genocidi ed esecuzioni di massa. Il rapporto continua con il denunciare decapitazioni, crocifissioni di bambini e sepolture di bambino vivi, cose che a leggere fanno accapponare la pelle. Tutte queste barbarie non sono poco note; addirittura, il sedicente Stato islamico ha pubblicato un manuale, La situazione della Nigeria non è molto diversa: sono definite come altrettanto allarmanti le barbarie perpetrate verso deboli, indifesi e minori per mano dei miliziani di Boko Haram, Boko Haram, un gruppo terroristico di etnia kanuri, che opera per lo più nel Nord della Nigeria, e che recentemente ha avuto un collegamento e si è affiliato al sedicente Stato islamico,

La comunità internazionale non ha avuto una reazione all'altezza di quello che sta accadendo. Ci si è limitati a semplici manifestazioni di sdegno o poco più.

Bisogna fare in modo che le potenze regionali del Medio Oriente possano essere in grado di esercitare pressioni verso il sedicente Stato islamico, i suoi *partner* e i suoi alleati. Analogamente si si dovrà operare con la Nigeria settentrionale e gli Stati del Nord, che sono in grado di esercitare un certo condizionamento, riducendo il più possibile la capacità operativa di Boko Haram.

dare impulso ad iniziative che portino all'accertamento dei fatti - conosciamo qualcosa, ma non ancora tutto - attivando tutti gli strumenti di aiuto e di supporto dell'infanzia in quei territori. Vorremmo anche che il Governo potesse dotarsi di strumenti più opportuni per identificare i responsabili di questi crimini contro i minori, prevedendone la possibilità di un deferimento alla Corte penale internazionale. Abbiamo poi un obbligo morale nei confronti dei cristiani che vivono in quelle zone. Occorre - a nostro avviso - valutare anche l'opportunità di inserire nel nostro ordinamento il reato di tentato genocidio, in caso di massacro indiscriminato di minori appartenenti a minoranze religiose, da potersi contestare a soggetti fermati in territorio italiano, sospettati di aver partecipato a stragi commesse anche all'estero, di cui siano rimaste vittime persone con meno di diciotto anni, uccise deliberatamente in ragione della loro appartenenza ad una minoranza confessionale.

del cospicuo numero di violenze, soprusi e abusi perpetrati sui bambini o aventi come protagonisti i ragazzi di tutto il mondo.

Nel mese di febbraio 2015 il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia ha diffuso nuove informazioni relative ad alcune pratiche brutali che il sedicente stato islamico (ISIS) attua nei confronti di minori. Da tale rapporto si evince che i bambini iracheni vengono rapiti e successivamente venduti come schiavi del sesso ed altri vengono crocifissi o addirittura bruciati vivi. Altri minori vengono usati come *kamikaze*, in particolare bambini con disabilità, oppure vengono usati come scudi umani presso i siti obiettivi degli attacchi degli Stati Uniti. Tale fenomeno ha ormai raggiunto livelli rilevanti. In tutto questo c'è un tale grado di aberrazione, uno sconvolgente stato di sgomento per le culture liberali, democratiche, fondate sul rispetto dei principi, della

bagaglio di sensibilità elettorali e di conquiste civili. È uno *shock* per le nostre secolari certezze e per la tenuta del diritto che nei secoli si è fatto garanzia per i deboli, per i piccoli e per gli emarginati. Libertà individuali che sono irrinunciabili, inalienabili, da difendere sempre e valorizzare quotidianamente. Bisogna farlo per noi e per tutti i popoli del Pianeta; farlo e continuare a farlo come diritto alla libertà per i nostri ragazzi e per tutte le bambine e i bambini del mondo. Tornando all'Iraq, anche le milizie irachene che combattono l'ISIS utilizzano i minori come soldati. Le crudeltà ormai comunemente perpetrate dall'ISIS non contraddistinguono solamente il comportamento e le azioni dei jihadisti del cosiddetto califfato, ma stanno caratterizzando anche altri gruppi e organizzazioni terroristiche, come Boko Haram in Nigeria, responsabile di crimini efferati nei confronti delle persone più deboli e, quindi, anche dei bambini. La radicalizzazione terroristica trova la propria spinta, oltre che nel fondamentalismo religioso estremo, anche nell'accaparramento del potere soprattutto economico in zone ricche di risorse naturali, ma poverissime di redistribuzione di ricchezza e irriguardose della qualità della vita di quelle popolazioni.

impegna il Governo: a richiamare i *partner* europei ed internazionali al pieno rispetto della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia sottoscritta da tutti i Paesi membri dell'ONU ad esclusione di Somalia, Sud Sudan e Stati Uniti; ad invitare, in occasione del prossimo Consiglio europeo, tutti i Paesi membri alla creazione di un comitato europeo per la vigilanza per la vigilanza del pieno rispetto dei diritti dei minori; a coinvolgere le associazioni *non profìt* operanti nei territori al fine di creare dei canali di aiuto ed intervento per tentare di arginare tale fenomeno che offende la dignità umana. Infine, mettendo in campo iniziative diplomatiche a largo spettro e relazioni internazionali, impegna il Governo ad invitare i Paesi dove hanno sede le aziende anch'esse operanti nei territori afflitti dalle organizzazioni terroristiche

di questo Governo per quanto accade nei conflitti armati in Asia, Africa, Sudamerica, e a poche centinaia di chilometri da noi, nel Medio Oriente, e anche nella vicina Ucraina. Potremo parafrasare la domanda del patriarca dei cristiani di Baghdad Louis Raphael Sako, che chiede - rivolto agli Stati Uniti ed all'ONU - dove sono gli americani che hanno invaso l'Iraq, cambiato il regime e annunciato che avrebbero portato i diritti dell'uomo, la democrazia e la libertà; dov'è dov'è la libertà; dov'è la democrazia. E dice che ora bisogna mantenere questo grande progetto e permettere a tutti i cittadini dell'Iraq di vivere dignitosamente. Nella zona siriana e nelle zone tra Iraq e Turchia in particolare, la condizione drammatica dei civili vede nella sua fascia più debole, costituita principalmente da donne e bambini, la privazione di ogni forma di diritto: alle donne sono imposte regole di sottomissione e segregazione; vengono punite in caso di violazioni con lapidazioni o impiccagioni. Le bambine, già dall'età di tredici anni, devono obbligatoriamente seguire tutti i dettami imposti alle donne. Inoltre sono in preoccupante aumento i matrimoni obbligati di queste ultime con i combattenti dell'ISIS, oppure sono rivendute come schiave del sesso, quindi subendo ripetutamente abusi sessuali e psicologici pesantissimi. I bambini vengono addirittura crocefissi, sepolti vivi, abusati e usati anche con scopo bellico e sono spesso usati nelle prime file dei combattimenti e, frequentemente, trasformati in bambini-bomba: uno scenario dell'infanzia istituisce il Comitato sui diritti dell'infanzia allo scopo di esaminare i progressi, compiuti dagli Stati parti, nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato. Il Comitato ONU può e deve chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione, pur nella consapevolezza che non ci possono essere soluzioni rapide per quella che appare essere una sfida generazionale, che deve essere contrastata con volontà politica, con risorse economiche e una disponibilità a sfidare le idee e gli atteggiamenti che stanno guidando l'espansione di questo fenomeno. l'osservazione passiva di questo Governo renda l'Italia complice. Il califfato continua ad espandersi mostrando di aver compreso la lezione della cosiddetta Primavera araba, facendo proprie quelle tecniche di comunicazione di avanguardia quali l'uso dei canali *social*, di video e *magazine* promozionali. In questa scia di terrorismo mediatico, si è inserito anche il gruppo nigeriano Boko Haram, che utilizza un canale multimediale attraverso il quale vengono mostrati immagini e filmati di minori impiegati in pratiche di addestramento militare. I *report* ONU evidenziano una situazione, sotto il profilo umanitario e della tutela dei diritti dell'uomo, nettamente critica e preoccupante. I bambini, i cristiani, fratelli mussulmani, l'ambiente, l'arte e la storia, anche quando risultano essere inoffensivi, sono visti e trattati con lo scopo di eliminare qualsiasi sfumatura di dignità umana, religiosa, culturale e artistica diversa da quella portata in esempio dalle milizie islamiche. Tutto ciò si traduce in crimini contro l'umanità, quali la riduzione in schiavitù, lo stupro e le violenze sessuali o di ogni altra natura, lo sfruttamento sotto ogni profilo possibile e la limitazione di tutte quelle libertà, intellettuali e materiali, innegabili per l'uomo e riconosciute oramai da anni dalla comunità internazionale. Il Comitato ONU sollecita, ad esempio - ed esorta lo Stato iracheno - a mantenere gli obblighi internazionali basati sul dovere della tutela dei diritti umani all'interno del Paese in ogni momento e ad adottare misure urgenti per fermare le violenze sui civili e contro i bambini. Inoltre si esorta ad istituire, oltre l'Alto commissariato per i diritti umani dell'Iraq, una sezione specializzata nella difesa e tutela dei minori. Si evidenzia, fra l'altro, l'importanza di attuare, celermente e senza indugi, leggi ferree contro le discriminazioni estreme di genere che colpiscono le donne fin dalle prime fasi della loro vita, esponendole con frequenza a violenze domestiche, abusi sessuali nonché psicologici. Il Comitato ONU esorta lo Stato a prendere tutte le misure necessarie per salvarli ed assicurare i responsabili alla giustizia, nonché a fornire assistenza ai bambini liberati o salvati dalla schiavitù o dal sequestro. Rispetto alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2015, ricordo una serie di azioni di stimolo ai Paesi *partner* che toccano vari aspetti che saranno parte anche delle nostre richieste di impegno al Governo: ad esempio una dura presa di posizione contro gli abusi commessi dall'ISIS nei confronti dei minori, mantenendo separate le azioni umanitarie da quelle militari e di antiterrorismo, cercando di rispettare il più possibile il diritto umanitario internazionale. Si chiede agli Stati membri di affrontare con urgenza la grave situazione delle donne e delle ragazze in Iraq e in Siria, dove subiscono pesanti soprusi i quali necessiterebbero di un'adeguata assistenza medico-psicologica oltre che di assistenza finanziaria. Si invitano le agenzie umanitarie internazionali attive in Iraq e in Siria, comprese le agenzie delle Nazioni Unite, ad aumentare la fornitura di servizi medici e di consulenza, tra cui l'assistenza e le cure psicologiche, oltre che a garantire un accesso all'istruzione. appoggia, infine, la richiesta, inoltrata dal Consiglio dei diritti umani all'ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, di inviare con urgenza una missione in Iraq per indagare sugli abusi e sulle violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani commessi dall'ISIS e dai gruppi terroristici associati. Affrontare una politica di tutela dei minori in quei luoghi significa affrontare anche il tema degli interessi dei cittadini cosiddetti occidentali, i quali ultimi ricevono indirettamente giovamento dall'azione delle compagnie multinazionali che ad esempio, in Nigeria, ricavano profitto dall'estrazione delle materie prime. materie prime. Dal delta del Niger e dalle *royalty* delle compagnie petrolifere dipende l'80 per cento delle entrate dello Stato nigeriano. Questo enorme flusso di denaro, unito alla pratica degli eserciti privati in difesa degli interessi delle compagnie, ha scatenato la violenza a tutti i livelli e i minori sono le prime, ma non le uniche vittime di questa ingerenza indebita. Va quindi riconosciuta una responsabilità occidentale dalla quale deriva l'obbligo di agire nella protezione dell'ambiente, delle risorse e quindi degli uomini, delle donne e dei bambini, data l'assenza di politiche specifiche per la tutela dei minori, delle donne o degli anziani in ambiti di guerra. Questo contesto deve impegnare il Governo, attraverso le organizzazioni internazionali che devono coinvolgere gli amici mussulmani moderati, che ricordiamo essere 1.600 milioni, a farsi promotore in sede europea delle conclusioni tratte dall'ONU attraverso la piena attuazione delle risoluzioni e dei rapporti citati, rivolti anche verso organizzazioni internazionali, ad elaborare strategie di intervento che vadano oltre l'intervento armato per contrastare i gruppi jihadisti nelle loro azioni a danno dei minori e delle donne, soprattutto per quanto riguarda la loro caratteristica di reclutamento giovanile mediante uso specifico di *media* e *social network,* a coinvolgere i *partner* internazionali nell'attuazione di un codice di comportamento, per le compagnie multinazionali che investono in Paesi con istituzioni democratiche instabili (proprio come la Nigeria), che preveda anche costanti informazioni sulle attività svolte, con particolare attenzione ai gruppi locali che esercitano mansioni di sorveglianza per le strutture e gli impianti. ad avviare una politica di cooperazione con il Governo nigeriano e con l'Onu volta a migliorare le condizioni sanitarie e di accesso alla scolarizzazione, soprattutto per i minori, attraverso un aumento costante delle *royalty* destinate a tale scopo e riscosse dai Paesi cooperanti nella percentuale spettante ai progetti di pacificazione e tutela dei minori, a verificare se attraverso la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa internazionale sia possibile agevolare nei casi di orfani di età inferiore ai tre anni, anche con disabilità lievi ed emendabili per motivi sanitari, l'adozione internazionale presso i tribunali per i minori per collegare le domande di adozione degli italiani, evitando così ulteriori violenze e ridando loro una famiglia.

Signora Presidente, il tema è quello che ha caratterizzato le mozioni illustrate dai colleghi che mi hanno preceduto e su cui siamo tenuti a mantenere siamo tenuti a mantenere un riflettore costantemente acceso. Ha ragione il collega Lucidi: in una parte del mondo si stanno perpetrando delle violenze, delle crudeltà, degli atti contro i diritti umani universalmente riconosciuti non soltanto dalle nostre Costituzioni domestiche, ma anche dell'Unione europea, di cui siamo parte integrante, e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ha fatto sì che il mondo

grazie a un meccanismo di tutela congiunta, inviolabile ed invalicabile, dei diritti umani fondamentali. Diritti umani che,

che c'è una parte del mondo che non possiamo più frequentare e conoscere perché è nelle mani di un integralismo islamista e di un esorcismo terroristico che ci impedisce di pensarla come una porzione di mondo caratterizzata da presupposti,

terrorismo, il quale, partendo dal Continente africano - e lo abbiamo visto, ahimè, attraverso episodi drammatici che non c'è bisogno di ricordare perché purtroppo sono stampati come un film nelle mente di tutti noi penetrano in Europa, nel mondo occidentale, a Bruxelles, a Parigi, a Madrid. Abbiamo, ahimè, un *cahier de doléances* e una categoria di sofferenze, disastri, crimini terroristici, che tendono ad essere in costante aumento. Tutto questo purtroppo ha un punto di partenza: il cancro del terrorismo islamista, l'ISIS, o Daesh che dir si voglia,

terroristico, di integralismo religioso islamista, ma con una vocazione e un progetto anche di carattere politico economico, che opera in Nigeria, attraverso l'agglomerato di movimenti sunniti, salafiti, wahabiti che, partendo da un apparente comune denominatore religioso, ambiscono alla conquista del mondo occidentale. Purtroppo l'abbiamo visto, perché, ahimè, uno dei tagliagole che abbiamo trovato tra i sodali dell'attentatore di Bruxelles, Salah Abdeslam, era proprio un nigeriano di Boko Haram.

nazionali, europei e mondiali, è lo sfruttamento indegno e inverecondo, da pornografia del dolore, della categoria più debole di tutte, quella dei bambini, dei minori. esistono dei campi di addestramento in Siria e in Iraq dove Daesh è diventato, come dicevo prima, un cancro o una malattia virale. Non saprei quale delle due patologie indicare come più adeguata, perché sono entrambe attagliate ad una forza che vuole distruggere il mondo attraverso il riflesso

costrette ad omicidi per entrare in schiavitù all'interno di queste organizzazioni criminali. Voi sapete che bambini dai sei ai dieci anni sono costretti a sparare, ad uccidere,

formati e diventano loro stessi formatori ancora minorenni. Proprio perché si utilizza la psiche infantile e la si strumentalizza, diventano i *killer* più spietati e incomunicabili. Tutto questo purtroppo caratterizza un sistema che ha visto in Boko Haram e nel Niger una delle punte più urgenti.

benissimo le dichiarazioni di intenti, le promozioni di sistema, ma ora come non mai, ora che è stato scalfito un movimento come Boko Haram, che rappresenta un esempio drammaticamente negativo per il terrorismo islamista internazionale, proprio in questo momento che li abbiamo indeboliti dobbiamo infliggere loro il colpo finale e definitivo.

trasparente del flusso di finanziamenti che arrivano (il famoso *money transfer* al contrario) nei nostri Paesi proprio per finanziare il terrorismo internazionale *in loco*, qui dove diventa più pericoloso. Tutto ciò deve essere reso tracciabile, visibile, contrastato e contenuto anche anche attraverso strumenti informatici che siamo in grado di contenere, controllare e censurare (colleghi, quando necessario dobbiamo usare anche questa espressione). Naturalmente chiediamo - lo abbiamo già fatto con altre mozioni e lo ribadiamo ora - che vengano intraprese operazioni di *intelligence* internazionale per identificare gli autori di questi crimini efferati e che ancora una volta si dia luogo a delle triangolazioni, a tavoli multilaterali internazionali in cui siedano l'Europa, l'Organizzazione delle Nazioni Unite e gli Stati africani, che aiutino a contrastare l'integralismo islamico, che si organizzino azioni positive a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, non solamente attraverso attività di volontariato, ma anche tramite azioni legislative da riflettersi sulle singole normative nazionali, che garantiscano una tutela dei minori sacrificati dal sistema del terrorismo internazionale.

acuisce gravemente la situazione, determinando ripetuti spostamenti di popolazione tra i due confini e verso il Kurdistan iracheno. Metà della popolazione siriana ha abbandonato le proprie case: i rifugiati sono stimati in circa 4 milioni, mentre gli sfollati all'interno del Paese sono circa 8 milioni. L'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari stima che il numero di persone in situazioni di bisogno di assistenza sia in aumento e corrisponda a più di 12 milioni di persone, un terzo delle quali vive in zone che sono difficilmente raggiungibili dagli aiuti internazionali. Siamo di fronte ad una delle più gravi crisi umanitarie al mondo, con oltre 5 milioni di bambini e di adolescenti coinvolti. E ai bambini siriani ai bambini siriani rifugiati nei Paesi limitrofi si aggiungono i bambini iracheni vittime del conflitto in Iraq. Tra l'altro, i diversi rapporti internazionali, dal rapporto della Commissione per i diritti del bambino delle Nazioni Unite del febbraio 2015 al rapporto annuale sulla situazione dei minori in zone di guerra, presentato dal Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, ci confermano che i conflitti attuali si caratterizzano per un totale disinteresse per la protezione dei civili in generale, con una particolare violenza nei confronti dei bambini. le parti in conflitto hanno ripetutamente violato il diritto internazionale umanitario ed hanno commesso altre gravi violazioni ed abusi dei diritti umani. il dramma che si trovano a vivere i minori negli scenari di guerra ha assunto davvero proporzioni che possiamo definire apocalittiche, tant'è che con sempre maggiore frequenza vengono denunciati casi di esecuzione di massa di bambini, con decapitazione, crocifissione, fino a sepoltura di bambini vivi. una situazione che definire agghiacciante è dir poco. A tutto questo si aggiunge il dramma dei bambini soldato, addestrati a combattere sin da piccoli, spesso usati come scudi umani o come *kamikaze*, oppure impegnati nella fabbricazione di ordigni esplosivi, per arrivare fino alla pratica della schiavitù sessuale, che colpisce donne e bambini. Al dramma siriano si aggiungono i drammatici aggiornamenti degli attacchi del gruppo terrorista di Boko Haram, attivo nel Nord della Nigeria e responsabile di atroci violenze a danno di civili e di attacchi suicidi messi in pratica utilizzando sempre più spesso minori, per lo più bambine. Basti ricordare la strage compiuta all'inizio dello scorso anno, nel gennaio 2015, con la stima prodotta da Amnesty International, che parla di circa 2.000 vittime. E stragi come quelle continuano ancora nel 2016.

naturalmente nei Paesi limitrofi e una parte sostanziale anche in Italia; si tratta di un numero certamente destinato ad aumentare in modo corposo nel 2016: è una delle più grandi popolazioni di rifugiati provenienti da un unico conflitto che si sia registrata negli ultimi anni. Possiamo dire che siamo di fronte al più grande esodo della nostra era, che coinvolge purtroppo in gran numero proprio i bambini. Venendo a noi, le stime di Save the Children dicono che il 40 per cento dei migranti arrivati in Grecia nel mese di febbraio di quest'anno sono minori. L'altro elemento di cui dobbiamo tenere conto è che i dati del Ministero dimostrano che i minori non accompagnati arrivati in Italia al 31 dicembre 2015 ammontano a circa 11.920, con un aumento del 13 per cento rispetto al 2014. Significativo e preoccupante, oltre a questo grande numero di bambini non accompagnati, è il dato relativo ai minori scomparsi: 6.150 bambini scomparsi dalle comunità di accoglienza.

il timore, forse anche la certezza, è che una parte consistente di loro sia caduta nelle mani di organizzazioni criminali e di trafficanti di esseri umani. Si parla, quindi, di sfruttamento sessuale, lavoro nero, addirittura commercio di organi. Abbiamo tenuto conto di questa

riconoscendo il lavoro importante che il Governo sta facendo, impegna il Governo a continuare a sostenere, in sede sia europea, sia internazionale, anche per il tramite di organizzazioni internazionali, una forte azione strategica, anche attraverso il ricorso a corridoi umanitari. Il tema, infatti, è portare soccorsi internazionali, ma anche permettere alle persone di uscire da quei Paesi e mettersi Questo, naturalmente, in favore di tutta la popolazione civile, ma - ripeto - i dati sui minori ci dicono che ci deve essere, così come chiedono le convenzioni internazionali, un'attenzione particolare sui minori che, sia per le violenze subite che per la loro piccola età, sono i più colpiti. Contemporaneamente, chiediamo di assicurare la protezione dei minori e che questo punto sia al centro di ogni risposta europea sulla crisi dei rifugiati. Questo anche per rafforzare e sostenente l'azione

il Governo anche a ricorrere all'affido familiare. Certamente c'è un tema di comunità e di accoglienza, ma crediamo che questo sia un punto importante, perché l'affido familiare è lo strumento attraverso il quale il nostro Paese oltre a garantire il rifugio ai minori non accompagnati e che sono in fuga dagli orrori del conflitto, anche a permettere la rottura di quei vincoli con gli ambienti jihadisti, nonché con le forme di reclutamento connesse.

sollecitando, ancora una volta, come è stato poc'anzi detto dalla senatrice Mattesini, l'intervento del nostro Governo in merito alla predisposizione dei corridoi umanitari per le popolazioni civili dilaniate dalle atrocità dei conflitti in corso nei territori occupati dall'ISIS e da Boko Haram. Poco meno di un mese fa uno dei più affermati storici italiani, Marco Impagliazzo, ha scritto per «Avvenire» un editoriale davvero illuminante. L'articolo si intitolava «Non rifare la cortina». Impagliazzo ammoniva il Vecchio continente sull'evenienza che la risposta migliore, o almeno una di quelle possibili, alla crisi dei profughi e dei rifugiati potesse rinvenirsi in politiche nazionaliste di arroccamento e di chiusura. In sintesi, l'ammonimento, richiamando le famose parole di Winston Churchill, si riferiva all'idea di non cedere alle tentazioni e alle spinte populiste volte a rispondere alle criticità crescenti con l'Europa dei muri e delle barriere, dei fili spinati e dei controlli spietati. L'obiettivo era ricordare che vi sono forze politiche che spingono alla creazione di una nuova cortina di ferro che rischia di essere calata ancora sull'Europa, tralasciando tutti quegli ideali e obiettivi che sono il fulcro dei principi e dei diritti su cui si fonda il sistema democratico del nostro Paese e dell'intera comunità europea: pace, legalità e solidarietà. Finora l'Italia si è dimostrata un Paese accogliente e solidale verso chi aveva e ha bisogno d'aiuto e assistenza, *in primis* quelle nostre Regioni maggiormente esposte ai flussi migratori. Detto questo, non possiamo però certamente tralasciare i numeri drammatici, testé detti, con i quali ci si confronta ogni giorno e che ci riportano drammaticamente alla realtà di oltre 3.500 uomini, donne e bambini (sono oltre 800 questi ultimi) annegati nel mar Mediterraneo nel 2015. memoria - abbiamo approvato in Senato la legge istitutiva della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. La legge contiene due priorità: conservare e rinnovare la memoria delle vittime e - soprattutto - all'interno delle scuole e in riferimento alle più giovani generazioni, formare l'opinione pubblica alla solidarietà nei confronti dei migranti e al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo. Insomma, occorre lavorare insieme a tutta la comunità per creare una realtà di integrazione e accoglienza. Se i cardini del nostro sistema di accoglienza si fondano quindi su concetti basilari quali l'inclusività e l'integrazione, la solidarietà e la speranza, l'accoglienza e l'uguaglianza, il diritto alla vita e alla salute, bisogna allora attivare e sostenere ogni iniziativa utile a dare alle istituzioni nazionali e internazionali quell'afflato umanitario senza cui la nostra identità, nazionale e comunitaria, è svuotata di ogni significato. Il progetto pilota sostenuto dalla Comunità di sant'Egidio, dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia e dalla Tavola valdese che, nel marzo scorso, ha permesso a 97 profughi di origine siriana di arrivare in Italia dal Libano, è stato un simbolo concreto di come poter intervenire in via preventiva, salvare vite umane ed evitare i cosiddetti viaggi della morte. La buona notizia, in un'epoca tragica per le migrazioni come quella che stiamo vivendo, è che entro la fine di aprile, cioè tra pochi giorni, ne giungeranno in Italia altri 150 tramite il percorso, sostenuto dall'Esecutivo, sicuro e umano dei corridoi umanitari, vero possibile punto di incontro tra istituzioni e società civile e strumento tangibile di integrazione. Finora l'esperienza dei corridoi umanitari è stata autofinanziata dalle organizzazioni italiane, cui va il plauso per l'azione svolta e spero vivamente si possano contagiare in quest'esperienza altri Paesi europei. un'esperienza in cui, però, *in primis* tutte le istituzioni italiane e la nostra società civile, devono credere per esportare un modello che può rappresentare un punto di svolta in tema di solidarietà, come ci ha ricordato qualche giorno fa anche il ministro Paolo Gentiloni.

ha aperto a Roma, dopo le sedi del Cairo e Atene, un centro di riabilitazione per i migranti vittime di tortura e trattamenti inumani, crudeli e degradanti. È di questi segnali che abbiamo bisogno, simboli palpabili di umanità e solidarietà che fioriscono nelle nostre comunità, magari lontani dai riflettori. migrante e del rifugiato papa Francesco ci ha ricordato come guardare a queste persone non significhi soffermarsi sulla condizione di regolarità o irregolarità, ma - soprattutto - vedere il lato umano di vite che vanno rispettate e tutelate nella loro più intima dignità. La solidarietà e la comprensione siano allora i cardini fondanti su cui la società italiana e quella europea, dal punto di vista istituzionale e sociale, possano ripartire.

contro l'odio e la bieca violenza fondamentalista, un vero sussulto di umanità possibile e assolutamente necessario. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, rappresentanti del Governo, con convinzione ho sottoscritto la mozione a prima firma Mattesini, che ringrazio, perché ritengo che l'attivazione di corridoi umanitari per minori e donne che fuggono da Paesi in guerra non sia più rinviabile. Non possiamo più tollerare le sistematiche violazioni dei diritti umani nei territori occupati da ISIS e Boko Haram, costantemente denunciate su più fronti e che io stessa avevo rappresentato all'Assemblea, nel febbraio 2014, tratteggiando con numeri e dati le condizioni dei bambini siriani. In quei territori ci sono donne appartenenti a minoranze etniche e religiose che vengono rapite, violentate e vendute come schiave, bambini sottratti con la forza alle loro famiglie per essere indottrinati alla guerra o utilizzati come scudi umani, bambine che subiscono destini indicibili. Sono contesti a dir poco allarmanti, che monitoriamo costantemente all'intero della Commissione diritti umani. Secondo l'UNICEF sono 5.600.000 i bambini siriani presenti ancora nella propria Nazione d'origine, devastata da una guerra che perdura dal 2011; mentre altri 2 milioni sono fuggiti nei Paesi confinanti. I bambini rappresentano, da soli, il 36 per cento dei migranti in fuga. I dati confermano, ancora una volta, come l'unica opzione sia quella di affrontare lunghi viaggi alla ricerca della pace e di una vita normale. È una scelta obbligata, che ha risvolti particolarmente drammatici. Solo nel 2015 sono stati 700 i

La foto di Aylan, che abbiamo già ricordato, è diventata immagine simbolo di un esodo disperato, un'icona potente, capace di smuovere le coscienze di buona parte dell'Europa sul tema dell'accoglienza. Ora però, non dobbiamo e non possiamo consentire che quello stesso scatto fotografico diventi il manifesto della nostra impotenza. Soltanto pochi giorni fa Amnesty International ha denunciato che le autorità turche da gennaio hanno iniziato a rimpatriare illegalmente migliaia di rifugiati siriani. Si tratta di uomini, donne (anche in gravidanza) e bambini. notizie gravi, emerse alla vigilia delle prime espulsioni previste dall'accordo Ue-Ankara, entrato in vigore lunedì scorso e su cui l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e le principali ONG hanno espresso molte preoccupazioni sia per la mancata tutele verso i migranti, sia riguardo alla detenzione dei richiedenti asilo. L'accordo, che è stato anche al centro dell'ultima audizione in Commissione per i diritti umani di ieri dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, che ha lasciato emergere una serie di criticità: *in primis* il rischio concreto che in Grecia - Paese che ha appena modificato la legislazione sulle richieste d'asilo - venga attuato un meccanismo di sommaria valutazione delle domande, che porti a una rapida dichiarazione di inammissibilità e, quindi, a una serie di trasferimenti forzati. È un dramma nel dramma che richiama l'Italia a esprimersi in merito al contenuto dell'accordo e noi parlamentari siamo in prima linea rispetto a queste responsabilità. situazioni meritano la massima attenzione, ma soprattutto risposte concrete. Rispetto ad altre realtà europee, il nostro Paese, pur con le criticità che conosciamo, ha mostrato la volontà di accogliere, grazie alla vasta rete di servizi offerti dalle istituzioni, dalle organizzazioni e dalle associazioni che operano sui territori. Ma non basta. Secondo l'ultimo «Rapporto sull'accoglienza

numeri disegnano una realtà inaccettabile, che va combattuta creando subito dei corridoi umanitari, perché almeno i minori non possano più finire nelle mani di trafficanti di essere umani e della criminalità organizzata.

La tratta degli esseri umani, fra i temi al centro del nostro impegno nella Commissione per i diritti umani, che a febbraio ha licenziato l'ultimo rapporto sui Centri di identificazione ed espulsione, riguarda molto da vicino anche le donne che fuggono dalle zone in cui imperversa Boko Haram. Si pensi che, secondo un rapporto dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), negli ultimi tre anni sono sbarcate in Italia quasi 7.000 donne nigeriane, 5.000 delle quali solo nel 2015. Fra queste ultime si contano circa un migliaio di minorenni. giovani e giovanissime che, nella maggior parte dei casi, non sanno neppure a quali rischi vanno incontro lasciando le loro terre, ingannate da false prospettive. Strappare questi corpi e queste anime alle organizzazioni criminali significa offrire un'accoglienza sicura per dare loro una vera speranza di una vita migliore. che, rispetto alla situazione siriana, in Nigeria si registra un cambio di passo nella reazione a Boko Haram con 11.600 ostaggi liberati nell'ultimo mese e programmi di recupero per questi ostaggi. In tal senso va anche la proposta di legge dell'onorevole Sandra Zampa, Vice Presidente della Commissione deputati, che prevede fondi certi per l'accoglienza, per evitare che debbano essere soltanto i Comuni a farsene carico. Si tratta di un provvedimento che pone anche più attenzione alla formazione, come pure ai percorsi di affido e supporto all'inserimento sociale. Molte buone pratiche si stanno attivando, ma non sono di sistema: persistono quindi le criticità nella fase di intercettazione del minore e di avviamento di percorsi di protezione.

attivare percorsi di potenziamento educativo nei Comuni e nei territori dove più forte è la presenza di minori stranieri di recente immigrazione, perché l'accoglienza possa andare di pari passo con l'integrazione e favorire l'inclusione. Per tutti questi motivi, sollecitiamo con forza il Governo affinché si impegni, a livello europeo e internazionale, per l'attivazione di corridoi umanitari e a garanzia di protezione dei minori, anche attraverso l'affido familiare, così come proposto nel dispositivo della mozione.

parte del paragrafo nel seguente modo: «nonché in particolare il reclutamento giovanile effettuato mediante uso specifico di media e *social network*, anche con mirate iniziative di contrasto all'estremismo violento».

capillare nel nostro Paese; 6) a continuare a sostenere il lavoro del Comitato per i diritti del fanciullo in modo da poter avere, in particolare attraverso i rapporti di monitoraggio periodico,

le seguenti «a continuare a sensibilizzare le compagnie multinazionali ed italiane affinché si attengano ai principi della responsabilità sociale d'impresa (CSR), tenendo - tra l'altro - anche conto degli UNICEF *children's rights and business principles*, inclusa la diffusione di ogni

«a continuare a promuovere negli opportuni contesti multilaterali l'adesione delle imprese agli strumenti internazionali esistenti in materia di *corporate social responsibility*» con le seguenti «a proseguire una politica di cooperazione con il Governo nigeriano, mediante gli organismi dell'Unione europea e dell'ONU, volta a migliorare le condizioni sanitarie e di accesso alla scolarizzazione, soprattutto per i minori»

e di Boko Haram; 6) a sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite a tutela dei minori e degli infanti vittime delle succitate violenze, eventualmente anche attraverso l'invio di una missione di pace delle Nazioni Unite, qualora ne ricorrano i presupposti;

siamo qui oggi a rilevare l'obbligo morale di richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sulle delicate tematiche trattate nella mozione presentata dal Gruppo dei Conservatori e Riformisti, insieme ad Non voglio soffermarmi sui molteplici trattati internazionali, tra i quali il più recente è la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, risalente al 2011, oppure la storica Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989, che testimoniano la formazione di una coscienza globale circa l'universalità e inviolabilità dei diritti dei più deboli e del diritto all'infanzia. Purtroppo, tristemente e sempre con maggior frequenza, siamo costretti ad assistere, impotenti, a reiterate a reiterate azioni che, in totale spregio della sacralità della vita - e particolarmente delle giovani vite - violano sistematicamente i diritti di milioni di bambini. L'infanzia viene regolarmente violata, purtroppo, e in forme diverse, in Cina, in Russia, in Thailandia, in Kazakistan, in Laos e Cambogia. Sono Stati ricchi di risorse naturali, dove

sono più gli affari che le libertà dei cittadini. Poi ci sono le guerre, con il Medio Oriente devastato dalle contrapposizioni cruente tra l'Islam più estremista e quello più moderato. Oppure c'è l'Africa, dove il dramma dei profughi - come ci è ben noto - arriva a toccare l'Italia, il Mediterraneo, l'Europa. Come sempre accade, sono le parti più deboli le donne, i bambini e i disabili - a essere più facilmente e brutalmente sfruttate, in Paesi dove l'intensità del conflitto armato ha raggiunto livelli di estrema violenza, con un impatto sproporzionato e intollerabile su queste categorie di persone. In Siria, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, ma anche in Somalia, Iraq, Afghanistan ed altri Paesi, migliaia di bambini sono reclutati, uccisi, mutilati, stuprati, indottrinati e obbligati a commettere atrocità. Ciò che più di tutto allarma sono i numeri. L'utilizzo dei bambini *kamikaze* è in aumento ed è in diminuzione la loro età. Le associazioni umanitarie parlano di 300.000 bambini bambini di età minore ai quattordici anni nei vari continenti. Da Boko Haram al Daesh, passando per le filiere qaediste in Pakistan, Somalia, Palestina, Yemen, cresce sempre più l'orrore dei bambini-kamikaze, arruolati a forza e usati come inconsapevoli strumenti di morte. lo Stato islamico non si fa scrupolo di addestrare, utilizzare e - in casi di necessità - anche di uccidere i bambini, reclutati dai predicatori dell'odio e attirati dal martirio offerto dalla *jihad.* Secondo quanto dichiarato al Consiglio di sicurezza dell'ONU dal rappresentante speciale delle Nazioni Unite per i minori nei conflitti armati - cito testualmente - «da gennaio 2014 in Iraq almeno 700 bambini sono stati uccisi o mutilati, vittime anche di esecuzioni Ex combattenti adolescenti hanno raccontato a ricercatori del gruppo per i diritti umani come i comandanti ribelli incoraggiavano i giovani a candidarsi per attentati suicidi. Ma non sono solo i gruppi jihadisti a usare bambini e adolescenti per azioni di guerra e di terrorismo. I minori combattono, purtroppo, nell'esercito regolare in Birmania, nella lotta armata contro le minoranze etniche, ma combattono anche in Ciad, nella Repubblica democratica del Congo, in Somalia, in Sudan, in Uganda e nello Yemen. Benché la maggior parte dei bambini-soldato siano maschi, anche le ragazzine rappresentano un numero significativo. Circa il 30 per cento delle forze armate mondiali che impiegano bambini-soldato hanno nelle proprie file delle bambine. Ci informano i *report* delle più autorevoli agenzie internazionali che le bambine vengono prima violentate, poi costrette a combattere o date in moglie

sono anche a capo di famiglie composte da mogli-bambine e i figli che nascono sono destinati ad ingrossare le fila dei combattenti. I bambini appena rapiti vengono costretti ad uccisioni anche di altri coetanei, così da farli sentire dei complici e legarli psicologicamente e indissolubilmente all'esercito. Nelle pieghe di queste drammatiche considerazioni sulle atrocità diventa impossibile non riconoscere un lucido e inquietante programma di radicalizzazione rivolto alle menti più giovani e fragili, perciò proiettato al futuro, al fine di forgiare la prossima generazione di terroristi jihadisti a più cruenti efferatezze. Sul fronte della campagna di espansione di Daesh, negli ultimi mesi il gruppo terroristico è stato molto attivo nella ricerca continua di reclute fresche, spesso servendosi della tecnologia e dei *social media*. Qui l'*information and communication technology* si fa involontaria complice e svela a noi uomini e donne del 2016, che confidiamo nella missione progressista delle ICT, tutta l'inadeguatezza e la fragilità dello sviluppo senza capacità di autocritica, privo di freni, all'assolutismo tecnologico. Laith Abbas, una giornalista, ex insegnante di Mosul e attivista per i diritti umani, ha dichiarato che la decisione dell'IS di «lavare il cervello ai bambini iracheni è l'ennesima tattica per trasformare la composizione religiosa della regione attraverso la paura e la coercizione». In uno stile molto simile a quello della Germania nazista, Daesh ha organizzato campi di internamento nelle aree sotto il suo controllo, per addestrare e rieducare migliaia di bambini iracheni e siriani di tutte le fedi. Questi figli dello Stato islamico sono diventati le nuove vittime di una aberrante forma di indottrinamento religioso di massa. Daesh non intende solo governare la regione, ma vuole che essa divenga teatro per la rappresentazione della sua ideologia, ideologia, servendosi della scoperta *pop* della ricerca occidentale, la più democratica in teoria: Internet. Per questo fine, vuole insediarsi nelle menti dei bambini, rimodellando il loro sistema di certezze nella uguaglianza degli esseri umani e smembrando e smembrando la loro bussola morale in accordo con il dogma. Recentemente, un autorevole rapporto medico sugli effetti dell'indottrinamento religioso su soggetti in giovane riferisce che le sofferenze fisiche e psichiche, imposte per rimodellare il sistema di credenze, produce effetti di lungo termine e causa nelle giovani vittime e causa nelle giovani vittime comportamenti asociali, violenza, psicosi, depressione e ritardo nell'apprendimento. E non potrebbe essere diversamente. Per tutti i motivi illustrati, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti considera proprio imprescindibile dovere morale tentare di sensibilizzare il Governo affinché si attivi per adottare le opportune misure, volte a salvaguardare il pieno rispetto degli inviolabili diritti dell'infanzia.

Io credo che intanto sarebbe necessario e urgente prima di tutto aprire corridoi umanitari sicuri, ma anche aiutare il Kurdistan iracheno, l'unica enclave in cui c'è una democrazia e in cui si rispettano i diritti umani.

intervengo solo per dichiarare il nostro voto a favore di tutte le mozioni presentate, nell'auspicio e nella speranza che un tema come questo possa essere trattato

una brevissima dichiarazione di voto sulla nostra posizione. Avevamo già valutato ogni singolo impegno di ciascuna mozione e avevamo individuato alcuni punti sui quali

fondamentalisti islamici e ceceni hanno ammazzato più di 300 persone, tra le quali 186 bambini. Non dobbiamo dimenticare le atrocità alle quali sono sottoposti i bambini: atrocità fisiche, crocifissioni, decapitazioni, bambini sepolti vivi e bambini *kamikaze*. Quindi, spero che ci sia l'impegno di tutti, da parte dei canali diplomatici e dell'ONU, di tutelare in termini effettivi i minori.

promosso questa discussione oggi in Senato sul tema della condizione dei bambini e degli adolescenti nei conflitti e nelle migrazioni e sulla necessità e urgenza di dare loro protezione e accoglienza. Dopo cinque anni di guerra in Siria siamo di fronte a una gravissima emergenza umanitaria. A causa del conflitto in Siria circa la metà della popolazione ha dovuto abbandonare le proprie case e il Paese è arretrato di quattro decenni. La conseguenza è che 7 milioni di bambini siriani sono ridotti in povertà e quasi 2 milioni e mezzo di loro hanno dovuto trovare rifugio nei Paesi vicini. Pensiamoci bene: tutti i bambini siriani sotto i cinque anni, 3,7 milioni di bambini, non hanno conosciuto da quando sono nati altro che la guerra con il suo carico di violenza, privazioni ed estrema precarietà. Secondo l'UNICEF, oggi più di 8,5 milioni di bambini all'interno della Siria e nelle regioni limitrofe hanno bisogno di assistenza immediata. Solo da questo Paese e solo nell'ultimo anno più di 15.000 minori hanno oltrepassato i confini in fuga non accompagnati e separati dai genitori. Si tratta di minori che si trovano, quindi, in una situazione - come si può comprendere - di grande vulnerabilità e soggetti a potenziali e gravissimi rischi. Voglio richiamare anche il dato - già ricordato da alcuni colleghi e colleghe - della situazione dei minori non accompagnati nel nostro Paese: sono circa 12.000 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto a quello dell'anno precedente. Circa la metà di questi minori fugge dalle strutture. Si tratta di un fenomeno in enorme crescita. Un terzo di questi viene ritrovato, ma degli altri non conosciamo la sorte. Una parte di loro riesce forse a raggiungere altri Paesi europei per ricongiungersi a parenti e amici. Vorrei sottolineare questo dato, perché penso sia un motivo in più e molto forte per chiedere, oggi più che mai, il superamento degli accordi di Dublino. È infatti evidente che questo superamento porterebbe a diminuire radicalmente i numeri di quanti fuggono per andare in altri Paesi europei. È evidente che ci troviamo di fronte a una palese e gravissima violazione dei diritti stabiliti nella Convenzione ONU. Il primo non rispettato è il diritto alla vita. Un altro diritto non rispettato è quello del bambino a essere protetto in caso di guerra, di guerra, protetto o protetta da ogni forma di maltrattamento, abuso o sfruttamento; ad avere protezioni speciali se si trova senza genitori; ad avere una protezione speciale e assistenza nel caso in cui sia un rifugiato, ad esempio se proviene da un Paese in guerra. L'Europa ha il dovere di aiutare questi bambini. Abbiamo il dovere morale oltre che politico di occuparci dei bambini e degli adolescenti che arrivano in Europa alla ricerca di pace e benessere, alla ricerca di una possibilità di futuro. A questa emergenza umanitaria alcuni Paesi europei hanno risposto con filo spinato, muri, treni chiusi, modalità di identificazione attraverso l'attribuzione di numeri, percosse perpetrate dalle stesse forze di polizia. Ciò che abbiamo visto e continuiamo a vedere sta accadendo in Europa e le immagini e le notizie che ci arrivano richiamano alla mente la tragedia del secondo conflitto mondiale, le deportazioni degli ebrei e i *lager*. Per questo ritengo che vadano utilizzate tutte le occasioni, come quella di oggi, per richiamare l'attenzione e denunciare questa situazione; per sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le istituzioni; per richiedere a tutti, a partire da noi stessi, il massimo impegno e responsabilità. Oggi è l'occasione per chiedere al nostro Governo di continuare ancora con più forza a esigere in sede europea e internazionale la protezione dell'infanzia e il rispetto della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Un punto va sottolineato a questo proposito: il compito e la responsabilità di accogliere e proteggere è di tutta l'Unione europea, non riguarda solo i singoli Paesi che si trovano di volta in volta interessati dalle rotte dell'esodo. La responsabilità è dell'intera collettività dell'Unione europea. È elemento costitutivo della nostra convivenza civile tutelare i bambini, la loro incolumità, la loro stessa dignità. Per questo nella nostra mozione abbiamo chiesto al Governo di continuare ad adoperarsi per una comune e condivisa posizione sulla gravissima situazione dell'infanzia e per richiamare l'urgenza di attivarsi, per affrontare con la massima decisione questa situazione presente nella nostra stessa Europa. La risoluzione più urgente è istituire dei corridoi umanitari che possano consentire l'arrivo, in modo sicuro e assistito, alle migliaia di bambini soli (i più vulnerabili) e anche a quelli con le proprie famiglie. Occorre mettere al centro di ogni risposta europea alla crisi dei rifugiati la protezione dei minori. Occorre poi sostenere tutte le iniziative, anche per il tramite delle organizzazioni internazionali, rivolte a garantire aiuto, assistenza e protezione ai minori. È necessario stabilire modalità e criteri per la presa in carico di queste persone, dei bambini innanzitutto, di questa infanzia che abbiamo l'obbligo e la responsabilità di tutelare e difendere. Dobbiamo in questo quadro continuare a incentivare, come ulteriore strumento di intervento, il ricorso all'istituto dell'affido familiare, che può consentire la protezione e favorire, oltre il necessario benessere, anche una positiva integrazione. Infine vorrei aggiungere, agli impegni e alle questioni poste nella mozione sottoscritta, oltre che da me, da numerose colleghe e colleghi del Partito Democratico, l'invito l'invito di procedere celermente all'approvazione del disegno di legge fermo alla Camera, che affronta e propone la revisione del sistema di protezione e presa in carico dei minorenni stranieri non accompagnati. Concludo, signor Presidente, dichiarando il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico alla mozione sottoscritta da numerose colleghe e colleghi del Partito Democratico Democratico stesso. Il nostro impegno continuerà su ogni iniziativa e azione rivolta ad assicurare ai bambini e agli adolescenti il diritto a vivere in sicurezza e in pace, il diritto alla loro stessa infanzia.

Non è bastato evidentemente l'appello di monsignor Moraglia, il patriarca di Venezia, ma neanche quello di monsignor Scola, che è il patriarca Sono state parole dure quelle che hanno usato questi due esimi rappresentanti del clero cattolico, con le quali hanno detto che l'urbanistica non può esistere come strumento di discriminazione e segregazione. Ciò che avviene oggi nel 2016 in Veneto assomiglia a ciò che avveniva nel 1500 con la nel 1500 con la nascita dei ghetti, e c'è voluto Napoleone per riuscire a chiarire che l'umanità deve convivere senza segregazione.

chi professa una religione diversa, come nel caso di quella islamica, a costruire le proprie chiese (quindi le moschee) tra i centri commerciali, nelle periferie e lontane dalle abitazioni. Va detto che questo risente di un'ignoranza palese. Sarebbe bastato chiedere alla Digos, ai Carabinieri, ai Servizi di sicurezza, per comprendere come oggi,

praticamente tutti, oggi predicano costantemente contro il terrorismo e a favore della pace e della convivenza rispettosa. Collaborano in maniera quotidiana e pregnante con le forze di polizia, si attivano nelle associazioni di volontariato e condividono lo spirito della Costituzione italiana, che è l'unico Vangelo laico che deve guidare l'azione legislativa sia nazionale che regionale. Altrove si annida il nemico che insieme vorremmo sconfiggere: in Internet, nelle periferie che si isolano dall'Islam pacifico,

Chi marginalizza oggi le moschee di fatto marginalizza il mondo islamico ed evidentemente fa il gioco di chi, invece, ha un interesse a far crescere l'odio reciproco e la volontà di segregazione.

Oggi chiediamo, pertanto, l'intervento del Governo italiano affinché si eriga il conflitto di competenza e il mancato rispetto della normativa europea sul paesaggio. Diciamo no allo scontro tra religioni in salsa veneta.

voluta dall'Organizzazione mondiale della sanità per celebrare il suo compleanno. Signor Presidente, colleghe e colleghi tutti, ribadire l'attenzione che a livello mondiale viene destinata in questa Giornata a un tema di particolare rilevanza, quale il diabete.

ritengo giusto le istituzioni debbano declinare per concentrare la propria azione legislativa sul versante normativo, ma anche regolamentare e regolatorio, al fine di dare maggiore impulso a quella che è una vera e propria pandemia,

L'impegno che si intende declinare in questa Giornata riguarda i temi della prevenzione, del rafforzamento delle cure, dell'attività di sorveglianza e delle attività inerenti la diagnosi precoce. In questo senso, mi permetto di evidenziare che proprio ieri presso l'Assemblea del Senato - analoga iniziativa è stata assunta anche alla Camera dei deputati - sono state presentate due mozioni *bipartisan* per impegnare il Governo a destinare una particolare attenzione a chi, nell'ambito della patologia diabetica, rappresenta una fascia di particolare fragilità e cioè i bambini. Il diabete a scuola, la necessità di garantire la continuità terapeutica e la somministrazione dei farmaci rappresentano una sfida che deve evidentemente impegnare anche quest'Assemblea. È questo il motivo per cui le

l'Organizzazione mondiale della sanità ha deciso che il protagonista della giornata mondiale della sanità oggi, 7 aprile 2016, sarà il diabete, una malattia silenziosa che nelle sue tipologie (tipo 1 e tipo 2) può creare seri problemi per la salute e la vita delle persone. Mi preme porre l'accento sul diabete di tipo 1 che rientra nella categoria delle malattie metaboliche a sfondo autoimmunitario e si manifesta prevalentemente nei bambini. La gestione del diabete di tipo 1, seppur è la stessa patologia da sempre, è cambiata drasticamente negli ultimi dieci anni. Dieci anni fa era una patologia che spesso veniva tenuta nascosta per paura di discriminazioni; la cura, cioè il dosaggio di insulina, veniva data dal medico e restava immutata per anni. Oggi questo mondo fortunatamente sta cambiando grazie innanzitutto ai medici e alle tante eccellenze italiane come il Meyer e il Bambin Gesù, ma grazie anche ai nuovi genitori aperti all'innovazione tecnologica

che, spesso, è un peso enorme per loro stessi e le loro famiglie. Oggi la terapia del diabete 1 è sempre più un complesso di azioni e valutazioni che ha un dinamismo veramente spinto, che si adatta a ogni specifico momento della giornata, in quanto il valore della glicemia non è influenzato solo da cosa si mangia - come avviene tipicamente nel diabete degli adulti (tipo 2), per i quali il rigore alimentare è molto spesso la principale cura ma dipende dagli stati emozionali, dall'attività fisica, dallo sviluppo ormonale. Ad oggi i microinfusori e i sensori glicemici dedicati sono prescrivibili in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, ma ci sono ancora dei limiti che dovrebbero essere rivisti. La ricerca e il progresso tecnologico possono fare moltissimo; il Governo e il Parlamento anche. Stiamo discutendo in questi giorni il codice degli appalti. Ci auguriamo che si possa andare oltre lo strumento delle gare e venga introdotto con chiarezza il criterio nell'aggiudicazione degli appalti della qualità e dell'appropriatezza terapeutica assistenziale per i dispositivi medici, perché ogni paziente ha il suo diabete. Si può fare molto per la qualità della vita dei bambini affetti da diabete 1, che hanno diritto a partecipare in modo inclusivo alla vita scolastica e sociale come tutti gli altri. Il Ministero della sanità e il MIUR con il Comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci a scuola hanno fatto dalla Società italiana di pediatria, dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Per questo motivo, insieme al senatore Lettieri e ad altri 81 senatori, abbiamo presentato la mozione di cui parlava il senatore D'Ambrosio ci auguriamo venga calendarizzata al più presto perché i genitori dei bambini affetti da questo tipo di diabete si aspettano da noi un provvedimento che renda la vita loro e dei propri figli più adeguata e normale.

negli ultimi mesi si stanno verificando dei fenomeni ripetuti e frequenti di microcriminalità, come furti in abitazione, che stanno destando molta preoccupazione in seno ai cittadini residenti. Questi ripetuti furti in abitazione da parte di bande di criminali hanno portato i gruppi di famiglie di queste tre contrade ad organizzarsi anche attraverso strumenti di comunicazione informatici per monitorare il territorio e lanciare allarmi in caso di ravvisata presenza di soggetti sospetti. Addirittura molte famiglie hanno stipulato dei contratti con il servizio di vigilanza urbana. I malviventi sono addirittura agevolati dalla mancanza di controllo del territorio da parte delle Forze dell'ordine nel *weekend* e nelle ore serali, in cui la caserma locale dei Carabinieri sostanzialmente sospende la propria attività. A parte un auspicato e opportuno intervento dell' amministrazione locale, del sindaco

dunque al ministro Alfano quali misure «intenda adottare per garantire il rispetto della proprietà privata e la sicurezza della cittadinanza a Città Sant'Angelo» e se, in particolare, intende potenziare l'organico della locale caserma dei Carabinieri, magari estendendone l'operatività

per discutere in modo efficace delle misure più appropriate per fronteggiare quella che a Città Sant'Angelo è una vera e propria emergenza in atto. *(Applausi del Signor Presidente, intervengo per pochissimi minuti, perché tengo molto a precisare a quest'Assemblea che il Resoconto stenografico della seduta di ieri, 6 aprile, non riporta per intero ciò che si è detto ieri. Ciò potrebbe aprire ad incomprensioni e giustificazioni per un'offesa ricevuta. Durante l'intervento della senatrice Ricchiuti, in cui chiedeva le dimissioni del conduttore televisivo Bruno Vespa e di tutto il gruppo dirigente RAI, ho espresso ad alta voce - forse anche dettata da una giornata abbastanza tesa - il mio punto di vista, che però non trovo nel Resoconto, dicendo chiaramente: «Chiedi le dimissioni di chi ha messo lì Vespa!». Mi ero curata, prima della chiusura della seduta dell'Assemblea, di richiedere ai funzionari stenografi di riportare tutto. Ciò perché la mia frase era comunque una reazione politica e non era un' offesa personale nei confronti della senatrice Ricchiuti. Vespa è un dipendente RAI e quindi ha un capo: Campo Dall'Orto e lo ha messo lì e lo ha imposto il Governo Renzi. La RAI è in mano al Governo Renzi; quindi, le responsabilità sono del Governo Renzi, che si avvale di ciambellani, come appunto aveva apostrofato la senatrice. La sua reazione - «Gallina, taci!» - rivoltami è stata chiaramente un'offesa alla mia persona. Il mio commento - lo ripeto - era un atto politico, rivolto a chi continua a dare ossigeno ad un sistema che si avvale di bravi servitori. La reazione offensiva della senatrice ha spostato tutto sul personale. Posso immaginare quanto male fa doversi rendere conto di far parte di una maggioranza sorretta da sistemi trasversali abbastanza imbarazzanti,

monodirezionale strisciante, che ha nome e cognome: potere. Detto ciò, invito a prendere atto di quanto ho dichiarato, affinché resti nei resoconti stenografici, almeno per quelli di oggi. Invito chi si scandalizza di tali giornalisti asserviti a guardare più in alto e ad evitare le offese gratuite. *(Applausi della

Questo è quanto oggi appare sulla prima pagina del «Corriere dello Sport». Sul caso del giorno interviene anche il presidente dell'Autorità

È normale che ciascuno di noi abbia una seconda vita sportiva o altre attrazioni al di là del lavoro, ma è anche doveroso mantenerle in quei canoni e in quei binari. Se l'altro giorno abbiamo dovuto sorbirci la ministra Boschi che a «Porta a Porta» ha paragonato l'importanza della mozione di sfiducia a quella di una partita di calcio del mercoledì sera, trovare il giorno dopo il principale protagonista dell'anticorruzione italiana che entra in questioni sportive francamente fa perdere il senso della realtà.

Lasciamo che sia Renzi ad apparire sul «Corriere dello Sport», ma mia dia retta presidente Cantone: ne stia lontano. Questo non fa bene al suo lavoro e neanche alla credibilità che tutti noi dobbiamo dare alle istituzioni.

Signora Presidente, il decreto-legge n. 149 del 2013 ha risposto alla necessità di superare il modello di finanziamento pubblico introdotto dalla legge n. 515 del 1993, che ha determinato il meccanismo dei rimborsi elettorali, stigmatizzato dall'interrogante per la mancanza di correlazione con le corrispondenti spese sostenute dalle formazioni politiche per la campagna elettorale. Il regime introdotto con la normativa in materia di abolizione del finanziamento pubblico diretto ha inoltre, con particolare riferimento alla trasparenza, disciplinato, all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 149 del 2013 l'obbligo di rendere accessibili le informazioni relative all'assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, nonché l'obbligo di pubblicare nei siti Internet gli statuti, il rendiconto di esercizio, completo di relazione sulla gestione e di nota integrativa, di relazione della società di revisione, nonché del verbale di approvazione del rendiconto stesso. Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati relativi ai finanziamenti e ai contributi erogati in favore dei partiti, al momento, esso resta assoggettato al rilascio del consenso, ai sensi della normativa sulla *privacy.* In proposito, l'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149, prevede gli obblighi di pubblicazione nel sito Internet ufficiale del Parlamento italiano, nonché nel sito Internet del partito politico, concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso. A tal fine, il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato, altresì, un provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale in data 6 marzo 2014, nel quale si precisa che, salvo i casi espressamente previsti dalla legge veda, ad esempio, l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013, come modificato dalla legge n. 13 del 2014, che prevede l'obbligo per i partiti di trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, nelle ipotesi ivi previste, l'elenco dei rispettivi sovventori), la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati relativi a soggetti che erogano finanziamenti o contributi in favore di partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico presuppongono il consenso degli interessati. Appare, pertanto, evidente che il decreto-legge n. 149 del 2013, convertito con modificazioni con la legge n. 13 del 2014, ha inteso smantellare il ventennale meccanismo dei rimborsi elettorali introdotto dalla legge n. 515 del 1993, seppure con la previsione di una fase transitoria prima dell'integrale attuazione della riforma, che opererà a completo regime nel 2017 (quando si saranno esauriti i pagamenti dei rimborsi elettorali). Nelle more della piena attuazione della riforma, le Camere hanno approvato la legge n. 175 del 2015 che modifica l'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 e interviene sulla funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Infatti, la Commissione di garanzia in questione, con comunicazione del 30 giugno 2015, rendeva noto di non essere in grado di proseguire il lavoro per carenza di personale e risorse. Quindi, la citata legge è finalizzata a rendere possibile il lavoro dell'organismo. con riguardo al preminente interesse della collettività alla trasparente ed economica gestione del denaro pubblico e al corretto funzionamento delle istituzioni, si ricorda che il decreto-legge n. 149 del 2013 ha introdotto, all'articolo 3, l'obbligo per i partiti di trasmettere il proprio statuto alla deputata Commissione di garanzia affinché questa ne effettui un controllo esteso ai contenuti sostanziali. Tale condizione ormai è stata ottemperata da quasi tutti i partiti rappresentati in Parlamento all'inizio della legislatura (come evidenziato dal sito della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che ha rilasciato le relative certificazioni di conformità), ma non dal movimento a cui appartiene l'interrogante. Questo elemento deve costituire oggetto di riflessione, perché proprio tale condizione ha permesso di compiere un ulteriore progresso in vista del raggiungimento di un livello alto di *accountability*. La posizione di partiti o movimenti che non si sottopongono a tale controllo ostacola il completamento di tale progresso, dato che impedisce la verifica e l'evidenza della conseguente responsabilità e della necessaria trasparenza delle regole sostanziali su cui si regge il partito o movimento che non ha ritenuto di depositare il proprio statuto. Tale risultato politico e istituzionale si pone in linea di continuità con il percorso annoso, e ancora non concluso, diretto alla completa attuazione all'articolo 49 della Costituzione, in merito al quale ogni parlamentare può esercitare la propria facoltà di iniziativa attraverso la presentazione di un progetto di legge. Per tali ragioni il Governo guarda con attenzione alle diverse proposte di legge presentate alle Camere, volte a definire in tal senso non solo il regime economico-finanziario del sistema dei partiti, ma anche lo *status* giuridico dei partiti stessi. Si tratta di un aspetto che, diversamente da quanto opinato da alcune parti politiche, risulta essere condizione imprescindibile dell'attuazione del dettato costituzionale.

pone un problema di coerenza rispetto all'interrogazione al Movimento 5 Stelle che finanziamenti pubblici non ne riceve e non ne vuole. Sono veramente costernato. Pensare di togliere i finanziamenti pubblici al Movimento 5 Stelle, caro Pizzetti, è come pensare di uccidere una talpa seppellendola viva. Noi stiamo bene così. Ben altro chiedevo e ben altro mi aspettavo in termini di coerenza dal Governo. Nel 2012, da sindaco di Firenze, Matteo Renzi

Queste sono le bugie del Governo che blandisce i cittadini con annunci ed elemosine e poi strizza l'occhio e stringe le mani alle *lobby* con regali miliardari. Lei, Sottosegretario, ci conferma che quelle somme sono state erogate, che i controlli non sono stati fatti e che la volontà dei cittadini è stata violentata, perché abbiamo votato chiaramente per abolire il finanziamento pubblico ai partiti e tale volontà è stata sovvertita solo pochi mesi dopo. Il finanziamento venne mascherato da rimborso elettorale, ma la Corte dei conti ha evidenziato il trucco: due miliardi di finanziamento, dei quali poco più di un terzo veramente documentato. Per parare il colpo la Corte dei conti oggi è sotto attacco. Evidentemente si vuole ridurre al silenzio chi indaga troppo e sul piano mediatico venne istituita una Commissione di garanzia per vigilare sui rendiconti dei partiti. Ma questa Commissione non vide mai assegnata - e lo ammette il Sottosegretario la quantità di risorse necessarie per lavorare e si trovò nell'impossibilità di svolgere il compito. Allora intervenne la sanatoria Boccadutri, con cui avete messo una cappa di omertà. Il Movimento 5 Stelle chiese almeno di dare più tempo alla Commissione, ma le casse avide dei partiti non volevano aspettare. Abbiamo proposto finanziamenti fossero erogati *sub iudice*, e cioè che venissero erogati ma, se poi emergevano irregolarità, potevano essere revocati. Nemmeno questo è stato accettato. Mentre i nostri imprenditori subiscono la mannaia inesorabile di Equitalia e quando chiedono credito devono prima dare garanzie, i partiti invece non devono darne nemmeno dopo. Allora, mentre i nostri imprenditori si spaccano la schiena e vengono sottoposti a un controllo spietato, quando entrano a gamba tesa i partiti si benda l'arbitro. Il Governo doveva mettere a disposizione dei cittadini quegli atti, e non subordinarli alla volontà dei partiti di renderli o meno disponibili. Doveva renderli integralmente disponibili: avrebbe trovato tantissime commissioni esaminatrici lavorato gratis, spontaneamente, per senso civico. Ma il Governo si fa beffe della trasparenza e con il solito acronimo inglese, FOIA (Freedom of information act), ha da poco lanciato un presunto atto sul diritto di informazione, ma tante e tali sono le condizioni e le eccezioni che tale atto si trasforma nella negazione di un diritto, in una presa in giro dove la pubblica amministrazione può negare le risposte semplicemente con il silenzio-diniego. E così è sufficiente buttare nel tritacarte la domanda per sottrarsi all'obbligo di rispondere. Eccolo il Governo. Viene in mente l'espressione: «Mi faccia causa» perché al cittadino rimane, come unica possibilità, rivolgersi al TAR, al buio, senza nemmeno sapere quali

al conflitto d'interessi della ministra Boschi e poi, recentemente, al caso del Ministro per lo sviluppo economico verso le *lobby* del petrolio. Le multinazionali scrivono gli emendamenti e il Governo li esegue, ma non è per questo che si chiama Esecutivo: dovrebbe eseguire la volontà del Parlamento. Noi siamo qui a chiedere che i dati sul finanziamento ai partiti siano integralmente messi a disposizione dei cittadini. Ma che ci possiamo aspettare da un Governo che, quando si chiede di discutere la sfiducia, dispone quando e come gli conviene? Ecco perché abbiamo un motivo in più, il 17 aprile, per votare sì al *referendum*.

Signora Presidente, l'interrogazione della senatrice Di Giorgi è volta a ottenere chiarimenti in merito a un concorso per l'assunzione di diverse figure professionali bandito dalla Regione Siciliana nel 2000, che ha dato adito a una molteplicità di ricorsi da parte degli interessati. Vorrei premettere che - come è noto - le competenze statali in materia di beni culturali siti nel territorio della Regione Sicilia sono esercitate dalla Regione stessa in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1975. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'arruolamento del personale tecnico impiegato nelle attività connesse alla tutela. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non ha pertanto alcuna competenza nella vicenda descritta nell'atto parlamentare della senatrice Si riferiscono tuttavia, in questa sede, per doveroso atto istituzionale nei confronti del Senato e degli interroganti, gli elementi informativi che, al riguardo, sono stati fomiti dal competente assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e del personale della Regione Siciliana. L'assessore regionale dei beni culturali, poco prima dell'entrata in vigore della legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10, ha bandito 19 concorsi per soli titoli, di cui 14 per 347 posti delle ex qualifiche di dirigente tecnico. Espletati i primi concorsi, con l'approvazione nel 2003 delle relative graduatorie, in considerazione della mutata disciplina applicabile alla dirigenza regionale per effetto della legge regionale n. 10 del 2000, si ritenne opportuno consultare l'ufficio legislativo e legale che, con parere n. 18740 del 5 novembre 2003, espresse l'avviso che il procedimento di inquadramento non poteva che rientrare «sotto il vigore della nuova normativa che a regime colloca nella categoria D - funzionari direttivi - gli assunti in possesso del diploma di laurea». Tale orientamento, pienamente condiviso dall'ex dipartimento regionale del personale della Presidenza della Regione, portò all'assunzione, con inquadramento in categoria D posizione economica 1, dei vincitori dei concorsi in oggetto. Il suddetto inquadramento ha determinato l'insorgere di un complesso contenzioso, che ha visto coinvolti circa 92 neoassunti e che si è sviluppato in tutti i gradi di giudizio, fino in Corte di cassazione. La sostanziale legittimità e correttezza del *modus operandi* seguito in ordine all'inquadramento nei nuovi ruoli regionali dei vincitori dei concorsi, banditi precedentemente alla soppressione dei ruoli tecnici, è oggi confermata dalla magistratura lavoristica, compresa la Corte di cassazione, che ad oggi ha esitato 18 sentenze favorevoli all'Amministrazione per 34 ricorrenti. Le conclusioni, dirimenti in materia, espresse dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 16728 del 2012 e confermate dalla sezione lavoro della medesima Corte nella sentenza 1403 del 2014, possono sintetizzarsi nei seguenti punti: il diritto del candidato vincitore ad assumere l'inquadramento previsto dal bando di concorso espletato dalla pubblica amministrazione. In regime di pubblico impiego privatizzato è subordinato alla permanenza, al momento dell'adozione del provvedimento di nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici, per i quali il bando era stato emesso, con la conseguenza che i vincitori assunti in esito ai concorsi *de quibus* non potevano pretendere la nomina in qualifica dirigenziale, messa a concorso,

quale disciplina esclusiva dell'inquadramento del personale già in servizio all'entrata in vigore della legge e non può trovare applicazione nei confronti dei dipendenti assunti in forza dei concorsi oggetto di controversia, assunti successivamente. Il successivo comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2000 va inteso quale strumento del legislatore finalizzato a evitare che fossero effettuate nuove assunzioni da parte della Regione fino al 31 con l'unica eccezione di quelle relative a concorsi indetti prima dell'entrata in vigore della legge, senza alcun riferimento al regime giuridico delle assunzioni medesime. per il personale non inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e per il personale direttivo, la determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l'individuazione dei profili professionali, distinti in relazione alla tipologia di prestazione lavorativa, è stata formalmente effettuata con gli atti di rilevanza generale, decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 2001 (e per altri aspetti con altro provvedimento),

l'Amministrazione per adempiere al suo obbligo di assunzione non poteva far altro che inserire il vincitore del concorso nella qualifica non dirigenziale di livello apicale (quella recante il grado D), non avendo essa la possibilità di creare una ulteriore qualifica, non essendone facoltizzata dalla legge» (pagina 13 della sentenza della Corte di cassazione n. 16728 del 2012). Sul punto della questione relativo alla disparità di trattamento tra un ridottissimo numero

inquadrati in categoria D/1, in esecuzione delle favorevoli decisioni della Corte di cassazione, si precisa che l'Amministrazione regionale siciliana ha sempre operato con il sostegno difensivo di tutte le avvocature distrettuali dello Stato delle diverse Province siciliane

funzionale messa a concorso, è la categoria D di nuova istituzione, per il cui accesso dall'esterno occorre il previo possesso del diploma di laurea. In tale categoria vanno inquadrati, a regime, i lavoratori addetti ad attività plurispecialistiche, con contenuto di tipo tecnico, gestionale e direttivo, e con risultati afferenti importanti e diversi processi produttivo-amministrativi, tra cui in particolare, come recitato nella relativa declaratoria, le figure professionali di psicologo, ingegnere, architetto, geologo cui sono assimilabili le figure inquadrate nel sistema previgente tra i dirigenti tecnici di cui ai bandi di concorso in oggetto. [DI

hanno vinto il concorso e si sono trovate, al momento dell'assunzione, a dover rinunciare alla precedente qualifica dirigenziale detenuta all'esterno. Certamente, è una scelta che hanno fatto, ma mai avrebbero potuto immaginare

non ha più garantito il livello per il quale avevano sperato di concorrere. Ringrazio il Governo per la risposta e per l'attenzione che mi ha dedicato.

l'interrogazione del senatore Molinari è volta a ottenere chiarimenti in merito agli interventi che si vogliono attuare per l'urgente salvaguardia del sito archeologico di Kaulon. Come è stato correttamente riferito nell'atto parlamentare, il sito dell'antica Kaulonia si trova nel Comune di Monasterace (RC), subito a Nord di Punta Stilo. Identificata da Paolo Orsi, al quale si devono i primi scavi, la piccola città Il tempio dorico fu ben presto acquisito al Demanio dello Stato, mentre la contermine fascia di abitato antico lungo il litorale è stata acquisita dopo il 2000 dal Comune di Monasterace. L'area statale e l'area comunale costituiscono il Parco archeologico dell'antica Kaulonia, il quale, insieme al Museo archeologico nazionale, ospitato in una sede di proprietà comunale, è stato consegnato nell'ottobre del 2015 dalla Soprintendenza archeologica della Calabria al Polo museale della Calabria. Il Parco non possiede strutture di servizio e non ospita personale fisso. La sua gestione in termini di manutenzione è mista. In occasione della grave mareggiata che investì la costa ionica calabrese tra i giorni 1° e 2 dicembre 2013, la Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria constatò l'aggravarsi delle condizioni di erosione del litorale prospiciente il Parco archeologico dell'antica Kaulonia, odierna Monasterace Marina, in particolare nelle zone dell'area sacra relativa al tempio dorico e del complesso termale, il cui famoso mosaico rende unico il sito di Monasterace nell'Italia meridionale La Soprintendenza chiese all'Università della Calabria, che già in precedenza si era occupata dello studio geologico dell'antica Kaulon e di altri siti magnogreci costieri calabresi, di eseguire un sopralluogo per valutare i danni arrecati dall'evento di burrasca e per proporre eventuali rimedi d'emergenza. L'esperta dell'Università, nella giornata dello stesso 2 dicembre 2013, eseguì il sopralluogo e contestualmente elaborò una relazione inviata alla Soprintendenza e all'allora commissario del Comune, con la quale, nel confermare la gravità della situazione, suggerì un primo intervento in emergenza, con la posa in opera di grossi blocchi a ridosso del deposito terrazzato su cui insiste l'antico insediamento. Negli stessi giorni la Soprintendenza chiese e ottenne dal Segretariato generale una somma di 300.000 euro per un primo intervento. Poiché le opere da eseguire esulavano dalle competenze della Soprintendenza, si chiese aiuto alla Provincia di Reggio Calabria, che con una spesa di 60.000 euro eseguì una barriera di protezione, ubicata sulla spiaggia davanti al tempio. La barriera della Provincia fu conclusa alla fine di gennaio 2014. Il 1° febbraio 2014 una nuova violentissima mareggiata investì la costa ionica, provocando nuovi gravi danni all'area archeologica. La barriera si dimostrò inefficace: una parte del muro di recinzione del tempio e un angolo del grande altare meridionale furono travolti dalla furia del mare. La direttrice del Museo con il suo personale recuperò tutto il materiale lapideo disperso dal mare e lo accantonò in Museo. Intanto si mise mano alla progettazione dell'intervento di urgenza di 300.000 euro; dopo studi meteo-marini e geologici e dopo aver consultato l'ufficio opere marittime del provveditorato alle opere pubbliche di Reggio Calabria, si decise di ricorrere a un progettista esterno. L'*iter* dell'intervento si è sviluppato nel corso del 2014, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 4 aprile 2015 e il collaudo si è concluso il 25 luglio 2015. Nel luglio del 2014, grazie a una rimodulazione di fondi, vennero concessi altri 700.000 euro dal Ministero per proseguire l'opera di protezione dell'intero fronte a mare del Parco archeologico, al fine di scongiurare danni da mareggiate al mosaico delle terme. Vorrei qui sottolineare che il famoso mosaico raffigurante draghi e delfini, coperto accuratamente dopo il restauro, non ha mai subito danni dalle mareggiate. Il progetto dell'intervento, finanziato con i 700.000 euro richiamati dal senatore Molinari, ha avuto un *iter* lungo e complesso ed è stato validato e approvato nel mese di agosto del 2015. Il Segretariato regionale, dopo la ricezione del progetto, ha chiesto alcune integrazioni, che hanno comportato ulteriore lavoro e l'impiego di ulteriore tempo. Con gli inizi del 2016 lo stesso Segretariato ha formalmente sollecitato l'indizione della Conferenza di servizi, che il 10 febbraio 2016 è stata convocata per il 9 marzo 2016. Preciso che il progetto prevede la realizzazione, in continuità con l'intervento conclusosi nell'aprile 2015, di un lieve rimodellamento del versante della duna costiera e l'inserimento di "gabbioni" in rete di acciaio riempiti di pietrame con pezzature diverse. All'interno dello stesso progetto è prevista un copertura a protezione dell'importante pavimento musivo. Purtroppo, nonostante alla Conferenza dei servizi del 9 marzo 2016 il progetto sia stato presentato come in fase definitiva, la fase attuale è quella di un progetto preliminare; il livello di definizione e di approfondimento progettuale dell'intervento presenta ancora delle lacune, quindi non è stato considerato adeguato ai criteri di selezione previsti dal programma PON cultura e sviluppo 2014-2020 e richiede ulteriori approfondimenti di tipo strutturale e idrogeologico. Si rende pertanto necessaria, anche alla luce dei pareri espressi in sede di Conferenza di servizi, una rapida rimodulazione del progetto che garantisca la messa in sicurezza della scarpata, rammento infatti che nel frattempo lo smottamento della duna dovuto all'azione del mare si è aggravato, discoprendo una sezione dalla quale emergono stratigrafie e strutture archeologiche, e la salvaguardia di quanto emerso; non più quindi solamente interventi di protezione dal mare ma una riprofilatura e rimodellamento dell'intero versante, previe adeguate operazioni di protezione delle preesistenze archeologiche e salva la definizione, in un momento successivo, di un progetto per il restauro dell'area archeologica. Vorrei rassicurare il senatore interrogante sul fatto che il nostro soprintendente sta provvedendo in tal senso, anche perché una maggior definizione del progetto potrà consentire la ricerca di nuove linee di finanziamento.

risposta, per onestà intellettuale, come in altre occasioni invece ho ricordato la difficoltà del Governo, alcune volte, a dare risposte al nostro lavoro di sindacato ispettivo. Spero che non sia vera la leggenda secondo cui risponde quando non ha responsabilità, anche perché in questo caso, invece, ha detto di essere molto attento al tema,

Signora Presidente, le interrogazioni cui si risponde vertono entrambe sul bando relativo ai Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale per il 2015, nello specifico sulla partecipazione del personale tecnico-amministrativo delle università ai gruppi di ricerca relativi ai singoli progetti. Si ricorda preliminarmente che il suddetto bando è stato emanato con il decreto direttoriale n. 2488 del 4 novembre 2015, il quale ha introdotto alcune significative novità rispetto alle precedenti procedure; Per la prima volta nella sua storia il PRIN ha aperto le porte, oltre che agli atenei e agli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche agli organismi di ricerca pubblici o privati, con ciò volendo favorire la più ampia concorrenza possibile tra i migliori studiosi e scienziati esistenti a livello nazionale. Inoltre, si darà completa attuazione alla portabilità dei progetti prevedendo che, nel caso di trasferimento del *principal investigator* o di un responsabile di unità da un ateneo o ente ad altro, il regolare svolgimento delle attività dovrà essere garantito semplicemente mediante accordo scritto tra i due atenei o enti. Ulteriore importante cambiamento riguarda le procedure di rendicontazione contabili a fine progetto, che potranno essere integrate, per le sole spese relative alla diffusione dei risultati, mediante produzione di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. Altra innovazione riguarda l'entità del finanziamento del Ministero, che non sarà più determinata in misura fissa, ma potrà variare di progetto in progetto. Sempre in rapporto al personale di ruolo, nel nuovo bando PRIN è prevista un'altra novità, consistente nella corresponsione, a scopo premiale, in favore dell'ateneo o ente sede di unità di ricerca dell'investitore principale, di una quota forfettaria per cento dello stipendio lordo annuo percepito dall'investitore principale al momento della presentazione del progetto, con conseguente sgravio dal calcolo dell'indicatore di sostenibilità finanziaria dell'ateneo, ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (ovvero dal calcolo del contingente di assunzione). Per quanto riguarda la valutazione dei progetti, questa avverrà in un'unica fase e sarà effettuata da tre comitati di selezione nominati dal MIUR e formati, per ciascun macrosettore, da esperti scientifici scelti dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca in base alla loro comprovata e specifica competenza. Come al solito, i comitati si avvarranno di revisori esterni anonimi (in numero di tre per ogni progetto), che opereranno in maniera indipendente, scelti dagli stessi organismi nell'ambito delle comunità scientifiche internazionali di riferimento. Tutta la procedura si svolgerà per via telematica, senza necessità alcuna di trasmissione e acquisizione di documentazione cartacea. Si comunica che alla scadenza del termine di presentazione, prorogato - lo ricordo - al 15 gennaio 2016, sono stati presentati 4.431 progetti e che, allo stato, è in corso la valutazione da parte dei citati comitati che si prevede potrà concludersi entro l'estate. Venendo allo specifico quesito posto dagli onorevoli interroganti, si precisa che il bando non ha impedito affatto l'inserimento nei gruppi di ricerca dei soggetti indicati all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (in particolare, per quanto qui interessa, del personale tecnico delle università). Molto più semplicemente, ai soli fini della valutazione scientifica da parte dei revisori, italiani o stranieri, individuati dal comitato di selezione del bando, la modulistica predisposta per la presentazione dei progetti ha richiesto che venissero esposti in un'apposita tabella soltanto cinque nominativi per ogni gruppo di ricerca, da scegliere, da parte del proponente del progetto, tra professori o ricercatori ritenuti maggiormente significativi dal punto di vista scientifico. Si è pervenuti a tale determinazione allo scopo di facilitare, in un'ottica di efficienza ed efficacia, il compito dei revisori che, in occasione di bandi precedenti ove tale limitazione non esisteva, si trovavano spesso di fronte a liste di decine e decine di persone per ogni unità di ricerca, senza che fosse chiaro il reale apporto e il peso scientifico di ciascuno di essi nella fase di realizzazione successiva dei progetti. Inoltre, a maggior chiarimento di quanto sopra esposto, con la FAQ n. 10 pubblicata sul sito dedicato al bando, si è precisato che il mancato inserimento nella tabella di cui sopra di un qualunque nominativo (ivi compresi professori o ricercatori) non precludeva in alcun caso la partecipazione al progetto. Proprio a tale scopo, si precisa altresì che il proponente del progetto, qualora lo ritenga opportuno, può fornire aggiuntive indicazioni in merito alla composizione e complementarità del gruppo di lavoro, inserendo ulteriori nominativi (oltre i cinque già previsti in tabella) nel testo del progetto stesso, in particolare nell'apposito paragrafo, denominato «Articolazione del progetto», con individuazione del ruolo delle singole unità operative e degli eventuali organismi di ricerca coinvolti in funzione degli obiettivi previsti

delle università italiane inquadrati come personale tecnico-amministrativo che potenzialmente guardavano con interesse all'ultimo bando PRIN. Si tratta di personale di alta o altissima qualificazione sia da un punto di vista formativo (hanno tutti la laurea e la maggior parte di loro ha anche un dottorato di ricerca o un diploma di specializzazione), sia da un punto di vista scientifico, in quanto si tratta di soggetti che partecipano all'attività di ricerca dell'università italiana, aggiungerei anche all'attività *tout court* di ricerca nel nostro Paese. Molti di essi hanno potuto ottenere, tra l'altro, l'abilitazione scientifica nazionale a posti di professore di prima e di seconda fascia. A fronte di questa preparazione, oggi il ruolo di questi veri e propri scienziati non è adeguatamente valorizzato essendo equiparati al personale amministrativo che, pur svolgendo un ruolo fondamentale per la vita dell'università del nostro Paese, sicuramente svolge mansioni e competenze molto diverse dai primi.

che la partecipazione di questo personale ai gruppi e ai progetti di ricerca è stato possibile soltanto di recente con la legge n. 240 del 2014. Negli ultimi due decenni, tra l'altro, in particolare nelle riforme che hanno riguardato l'università italiana, non si è considerata l'opportunità di una riqualificazione del ruolo del personale tecnico-amministrativo, anche con l'obiettivo di rendere più efficiente il sistema di ricerca universitario italiano. A oggi restano per questa categoria discriminazioni di fatto intollerabili. Apprezzo la sua risposta, ma ma quelle discriminazioni continuo a ritrovarle nell'ultimo bando PRIN e si traducono nel fatto, per esempio, che, per quanto in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, per questo personale è quasi impossibile, di fatto, essere chiamati a posti di professore, sia di prima che di seconda fascia, nonostante la legge n. 240. Per questi motivi penso che la questione che insieme agli altri firmatari abbiamo sollevato con questa interrogazione riguarda soltanto incidentalmente il bando PRIN. È arrivato il momento di superare queste discriminazioni, modificando l'attuale quadro normativo al fine di consentire a questo personale di essere inquadrato in un ruolo che possa valorizzarne le competenze. Penso, per esempio, al ruolo di tecnologo, previsto già oggi per tutti gli enti di ricerca pubblici del nostro Paese. A mio parere, a fronte di costi molto contenuti per queste modifiche, si otterrebbe, tra l'altro, la possibilità di incrementare nell'università il numero di risorse umane pienamente riconosciute come spendibili nelle attività didattiche e di ricerca.

per definire finalmente lo stato giuridico di ricercatore. Ovviamente, tifiamo per questa soluzione e per questo, signor Sottosegretario, mi auguro di poter contare sull'apporto del Ministro

Signora Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Toccafondi, perché, nel prendere atto che che il bando non prevede un'esplicita esclusione della tipologia del personale cui ci riferiamo nell'interrogazione, probabilmente si è determinata un'autoesclusione o, quantomeno, una una parte dei gruppi di progetto è stata indotta a escludere questa consistente fascia di collaboratori.

alla tenuta delle varie fasi progettuali, allo *start-up* del progetto,

del progetto in discussione. La verità è stata qui enunciata e, purtroppo, risale ad una mancata in merito alla qualifica e al ruolo del personale dei cosiddetti tecnici laureati, di cui ci siamo